al dettato costituzionale, a quello dell'articolo 119, introdotto dalla riforma del Titolo V del 2001, che, a distanza di otto anni, è ancora in larga parte disatteso. Finora il meccanismo dei rapporti finanziari tra il livello centrale e i livelli periferici è stato essenzialmente riconducibile al modello della finanza derivata, non essendo sufficienti le innovazioni introdotte in questi anni a favore dell'autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali a qualificare il sistema come una reale responsabilizzazione di tali enti nella gestione delle entrate e delle spese di competenza. Con il varo del federalismo fiscale abbiamo l'opportunità per l'intero Paese, dal Nord al Sud, di rendere la macchina pubblica più efficiente, sia ai livelli centrali che a quelli periferici. Nel dibattito politico si è in taluni casi parlato del disegno di legge n. 1117 come espressione dell'esigenza di una sola parte politica. Ritengo, invece, che con l'approvazione del testo in esame si introducano elementi significativi nel processo di riforma che il Governo e la maggioranza hanno avviato con risolutezza, procedendo notevolmente in tale cammino nel primo anno di legislatura (ricordo che proprio oggi cade il primo anno di legislatura). Nel modo in cui l'intendiamo, il federalismo fiscale non è un simbolo, una bandiera da agitare, ma uno strumento concreto per avvicinare l'azione delle pubbliche amministrazioni locali alle esigenze espresse dal territorio e dai cittadini, offrendo gli "attrezzi" per intervenire efficacemente. In tale quadro, il presente disegno di legge deve essere accostato alle altre iniziative messe in campo nell'ultimo anno come, ad esempio, il «disegno di legge Brunetta» - per rendere più efficace ed efficiente l'azione della pubblica amministrazione. Entrambi i provvedimenti muovono su piani diversi ma convergenti, nel senso della responsabilizzazione dell'iniziativa pubblica rispetto agli obiettivi del buon governo. Così come lo stesso federalismo fiscale potrà essere adeguatamente affiancato dal nuovo codice delle autonomie, che il Governo si accinge a predisporre, per una chiara e precisa definizione delle competenze e delle funzioni tra i diversi livelli di governo. Il presente disegno di legge ha avuto una genesi e un *iter* particolarmente complessi, che hanno però evidenziato come, pur nella legittima differenza di opinioni tra gli schieramenti, ci sia una diffusa consapevolezza in Parlamento e nell'intero sistema pubblico circa la necessità di dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione. In tal senso si può leggere il risultato del voto, espresso sia in quest'Aula in prima lettura, sia alla Camera, con l'astensione del principale Gruppo di opposizione, che fa seguito a un processo di dialogo e di condivisione che ha permesso di valorizzare le idee e le proposte provenienti da diverse parti politiche.

Il passaggio parlamentare alla Camera dei deputati ha consentito di introdurre ulteriori modifiche, che, a mio avviso, vanno nel senso di un complessivo miglioramento dell'impianto di delega. Mi soffermerò solamente su un aspetto, relativo al coinvolgimento dei livelli locali nel contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, prevedendo meccanismi di carattere premiale, così come testualmente recita il comma 2, lettera *d)*, dell'articolo 2. Tema, questo, ripreso anche dal nuovo articolo 26, introdotto dalla Camera, specificamente per il contrasto all'evasione fiscale, laddove si prevedono sia forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono Regioni, enti locali e Stato, sia forme premiali per Regioni ed enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Un passaggio che ritengo particolarmente significativo, perché indubbiamente segnala una corresponsabilizzazione delle amministrazioni regionali e locali in ordine non soltanto alla gestione della spesa, ma anche all'acquisizione dell'entrata, legata alla capacità fiscale di ogni territorio. Una responsabilizzazione che è fondamentale per un rapporto diretto tra elettori ed eletti, sulla base della trasparenza e della chiara definizione di risorse ed obiettivi, che viene ribadita in altre disposizioni, come quelle contenute nel comma *i)*, dell'articolo 2, laddove si prevede l'obbligo di pubblicare nei siti Internet i bilanci di Regioni ed enti locali, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese *pro capite*. Sarebbe sbagliato, a mio avviso, puntare sul federalismo fiscale come allo strumento per dare fiato ai bilanci dei Comuni o per tappare i troppi buchi di bilancio, spesso afflitti dalle alchimie della finanza creativa, come i derivati. Occorre invece comprendere che il federalismo va coniugato con autonomia e responsabilità, come appunto prevede il testo varato dal Governo. L'inefficienza complessiva delle strutture pubbliche è il più grande peso di cui si deve liberare l'Italia per diventare davvero un Paese "normale". Uno Stato che assorbe oltre la metà di quanto prodotto da tutti i cittadini appare autoreferenziale, cioè impegnato in gran parte a conservarsi immutato, estraneo quando non oppressivo verso le esigenze della società. Tramite il processo federalista, la responsabilità della spesa pubblica verrà decentrata, arrivando fino al livello più vicino possibile al cittadino a cui è destinata, che potrà così rendersi conto direttamente se quanto paga in termini di tasse è proporzionato a quanto riceve. Il fisco federale costituisce inoltre un'opportunità di riordino del complesso sistema di tassazione in vigore, frutto della sovrapposizione di iniziative diverse, che nel corso degli anni hanno determinato un intreccio di aliquote e addizionali che non contribuisce a un rapporto trasparente tra cittadino e amministrazione. All'ampia capacità di spesa decentrata deve dunque corrispondere un'altrettanto decentrata facoltà di tassazione, collegando specificamente il cespite soggetto a imposta con le funzioni che il livello di governo beneficiario della medesima è chiamato a svolgere. Oggi, con la prevalenza dei trasferimenti che dallo Stato ricadono a cascata su Regioni, Province e Comuni, è spesso praticata la tentazione di dare la responsabilità ad un altro livello, sia dello Stato nei confronti degli enti locali, che viceversa. Con il federalismo questi atteggiamenti di distorsione delle rispettive responsabilità non saranno più praticabili. Ogni amministratore sarà responsabilizzato davanti ai cittadini non solo per quello che fa o non fa, ma anche per il livello di tasse imposte, cosicché gli elettori, ad ogni turno elettorale, potranno valutare le realizzazioni e le tasse pagate e decidere se confermare o meno l'amministratore uscente. È un processo, in conclusione, che richiede anche una profonda maturazione dei cittadini, che devono abituarsi a fare il conto dei costi e benefici dei servizi pubblici. E per gli stessi amministratori di Regioni ed enti locali sarà lo stimolo per introdurre principi e metodi efficienti nella gestione delle risorse pubbliche. Oggi, per far funzionare la macchina burocratica, ci sono Regioni che spendono tre volte più di altre; basterebbe questo solo dato per avvalorare la tesi che un federalismo fiscale ben fondato, basato cioè sulla responsabilizzazione degli amministratori e una sana competizione tra territori, potrà consentire forti risparmi di spesa o una maggiore efficienza dei servizi.

Per rimettere in quadro i conti italiani, per arrivare alla media debito-PIL europea, pari a circa il 68

fila. È evidente a tutti che la situazione non si può risolvere con le finanziarie e con i piccoli aggiustamenti. Questa è la grande intuizione di Umberto Bossi: non è possibile sistemare i conti dello Stato con semplici aggiustamenti annuali. rifare tutto e rimettere tutto il sistema a regime con regole nuove e certe, quindi aggredire quegli 800 miliardi di uscita, perché non si fa niente con il piccolo aggiustamento annuale.

la responsabilizzazione degli amministratori locali, una forte riduzione della spesa pubblica e il contrasto all'evasione fiscale. Come? La responsabilizzazione degli amministratori locali tramite l'istituto - chiamiamolo così - del fallimento del politico: un politico che sfora e sbaglia semplicemente diventa ineleggibile; la riduzione della spesa pubblica con il passaggio dalla spesa storica ai costi standard; il contrasto all'evasione fiscale con il conflitto di interessi che si crea a livello locale, perché gli enti locali, trattenendo quote importanti di imposte, in particolare di IVA, avranno tutto l'interesse a stanare gli evasori per poter dare servizi migliori. Questi tre obiettivi alla fine vanno visti insieme

va da sé che la differenza va coperta diversamente: o riducendo l'inefficienza o recuperando evasione fiscale, altrimenti il sistema non tiene. tiene. Questo è il succo del discorso. Finalmente il federalismo fiscale dà un nuovo quadro di riferimento economico della redistribuzione di oneri e di risorse a tutto il sistema degli enti locali. Però giustamente guardiamo anche avanti. Il ministro Calderoli ha già illustrato i punti essenziali del riordino degli enti locali. riordino degli enti locali. Tale riordino è l'altra faccia della medaglia: mentre con il federalismo fiscale si mette a posto il quadro economico di riferimento, che già da sé automaticamente porta a un riordino del guazzabuglio - scusate il termine - presente nel sistema degli enti locali, è opportuno che si acceleri anche su questo L'articolo 114 della Costituzione, primo comma, dice semplicemente che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. Non ci sono comunità montane, consorzi, bacini imbriferi, ATO e compagnia cantante: l'elenco potrebbe continuare per pagine e pagine. Quindi va da sé che possiamo rottamare da subito tutti questi enti. Tutti e subito. Questa è una grande opportunità che abbiamo a Costituzione e a sistema normativo vigenti: la possibilità di ottenere un enorme risparmio e una semplificazione da portare avanti insieme al federalismo fiscale. Un secondo tema legato al riordino degli enti locali è quello delle Città metropolitane. Mi dilungo su questo tema specifico anche per non ripetere argomentazioni che stiamo già sviluppando un po' tutti. Fortunatamente - è un mio personale parere - le Città metropolitane non sono ancora partite, altrimenti ci troveremmo con un ulteriore livello locale, un ulteriore carrozzone da gestire nel sistema degli enti locali. Il dibattito che si sta aprendo sul ruolo delle Province può essere in quest'ottica un'opportunità. Quindi, perché non far diventare semplicemente queste Città metropolitane delle super Province quali le attuali, con le stesse regole di costituzione, magari con qualche funzione in più di area vasta, ma nient'altro, evitando di inventare l'acqua calda e di creare altra confusione, visto che ce n'è già a sufficienza,

che rivolgo per aprire uno spiraglio sul lavoro che ci aspetta domani. Siamo consapevoli che fin qui, grazie ai ministri Bossi e Calderoli, si è fatto un ottimo lavoro e sul federalismo fiscale siamo a posto, ma sappiamo che c'è ancora tanto da fare. Ci aspettiamo dall'opposizione lo stesso spirito collaborativo e costruttivo che c'è stato nell'approntamento del disegno del federalismo fiscale anche sul Codice delle autonomie. Siamo fiduciosi che ciò avvenga. *(Applausi

il disegno di legge sul federalismo fiscale giunge oggi alla fase conclusiva e all'approvazione, in seconda lettura, da parte del Senato, che lo aveva varato in prima lettura il 22 gennaio scorso. Siamo quindi in dirittura d'arrivo ed è legittimo esprimere la soddisfazione per un traguardo raggiunto con il concorso di tutto il Parlamento. Siamo consapevoli che questo è un momento storico della nostra Repubblica e lo dimostrano anche i numerosi interventi in quest'Aula in sede di approvazione conclusiva. Finalmente, in attuazione del dettato costituzionale, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono disporre di autonomia finanziaria per le entrate e per le spese. Ma per armonizzare questo principio fondamentale della nostra Costituzione c'è voluto un paziente lavoro di coordinamento legislativo tra la struttura amministrativa nazionale potremmo dire "piemontese" - che ha retto per 150 anni dall'Unità d'Italia e le diffuse esigenze di decentramento decisionale che hanno visto la significativa convergenza politica delle Regioni settentrionali con quelle del Mezzogiorno. Il federalismo in tal modo è in grado di promuovere lo sviluppo economico, ma anche la solidarietà sociale tra Nord e Sud. Il risultato più evidente è quello di una rinnovata coesione nazionale - che esalta le diversità - con l'effettivo esercizio dei diritti da parte dei cittadini italiani. Il gettito fiscale è oggi strettamente legato al territorio, in armonia con la Costituzione. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni dispongono di risorse finanziarie autonome potendo stabilire tributi in un rapporto diretto con i contribuenti residenti nel territorio. Ma la sperequazione tra Nord e Sud è fortunatamente scongiurata: viene, infatti, istituito un fondo perequativo a favore dei territori con minori capacità fiscali. In tale direzione vanno considerate le importanti modifiche apportate dalla Camera al testo che era già stato approvato dal Senato; esse consentono una puntuale attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. importante la modifica introdotta all'articolo 2, che si intitola «Oggetto e finalità» della riforma federalista e che individua gli strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30, 31 della Costituzione, con particolare riguardo alla formazione della famiglia. introduce un importante riconoscimento della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio (articolo 29), evidenzia il dovere ed il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio (articolo 30), e afferma che lo Stato deve agevolare con misure economiche e altre provvidenze

come vero ammortizzatore sociale e principale agente del *welfare*. La norma va, dunque, salutata con ottimismo, soprattutto perché dà il via ad una più ampia rivisitazione fiscale che pone al centro la famiglia e non il singolo individuo. In tal modo si va a correggere quella grossa sperequazione subita dalle famiglie numerose, soprattutto in termini di costi più che di benefici fiscali. In particolare, si apre la strada al quoziente familiare e, quindi, si apre una porta ad interventi più strutturali a favore della famiglia, soprattutto in un periodo di crisi economica globale. Un'altra importante novità - che voglio ricordare, anche se riguarda il primo passaggio al Senato - è stata la previsione di meccanismi premiali per gli enti che favoriscono l'occupazione e l'imprenditorialità femminile e la previsione del principio di pari opportunità. In particolare, l'ordine del giorno che prevede l'osservanza del principio di pari opportunità in un momento importante come sarà quello dell'emanazione dei decreti attuativi. Desidero di questo ringraziare il ministro Calderoli e il relatore, senatore Azzollini, perché in quella sede hanno recepito gli emendamenti a mia firma insieme a colleghe della maggioranza e dell'opposizione. In tal modo, il federalismo potrà correggere uno squilibrio che da troppo tempo pesa all'interno del sistema economico nazionale, penalizzando l'occupazione femminile. Va, inoltre, sottolineato che le enunciazioni innovative del federalismo fiscale assumono particolare rilievo anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica a livello nazionale. Per esempio, è previsto che le leggi regionali possano calibrare le accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, in rapporto ai cittadini residenti e alle imprese che abbiano sede legale e operativa nelle singole Regioni interessate. Sono inoltre previsti, in armonia con le norme comunitarie, interventi speciali in favore degli enti locali per garantire il loro sviluppo economico e sociale e per sopperire al deficit infrastrutturale, a una loro non ottimale collocazione geografica, ai diritti della persona, ai territori montani e alle isole minori. Sempre in tema di rapporti finanziari tra Stato e Regioni, assume rilievo la modifica introdotta dalla Camera, in base alla quale le Regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali. È anche questo un intervento sicuramente apprezzabile, perché l'IVA è un tributo più omogeneo, dato che il consumo non si differenzia, se non per i volumi, a livello territoriale. Abbandonare la strada dell'IRPEF, dunque, per concentrarci con maggiore attenzione sulle compartecipazioni all'IVA è uno sforzo importante.

obiettivi del Governo vi è quello di eliminare gradualmente questo tributo che ha creato solo scompensi nel sistema. Infatti, non è pensabile che un tributo incentrato sul valore della produzione non consenta la deduzione dei due principali fattori della produzione: il costo del lavoro e gli oneri finanziari. Il federalismo, inoltre, porterà una maggiore responsabilità per i cittadini, chiamati a dare il proprio voto alla gestione amministrativa. Ancora, è questo un altro punto che mi preme sottolineare, grazie al federalismo si avrà anche un'accelerazione della lotta all'evasione fiscale.

dell'Agenzia del territorio, dell'Agenzia delle entrate, volta a stabilire quali sono le discrasie e come mettere in comunicazione le banche dati. È infatti questo uno dei temi importanti che rappresenta uno dei punti di maggior rilevanza dell'intero provvedimento. Oggi l'ammontare dell'evasione fiscale in Italia è di circa 300 miliardi di euro di imponibile che vengono sottratti all'erario. Di questi, l'evasione di imposte dirette ammonta a 115 miliardi di euro, l'economia sommersa ammonta la criminalità organizzata sottrae 40 miliardi e altri 25 miliardi sono attribuibili a chi ha il secondo o terzo lavoro. Grazie al federalismo fiscale, dunque, si potrà realizzare una nuova cooperazione tra istituzioni, volta a combattere l'evasione stessa. avvicinando il destinatario del prelievo al soggetto che produce la ricchezza, sarà possibile assicurare maggiore trasparenza nel rapporto tra cittadini e istituzioni. Inoltre, il recupero delle imposte evase potrà permettere agli enti locali di finanziare i servizi forniti a livello decentrato. Già durante la prima lettura al Senato avevo proposto con un mio emendamento che fosse introdotto un sistema di incentivi che stimolassero le singole Regioni e gli enti locali a partecipare attivamente al recupero dell'evasione fiscale, prevedendo la possibilità per le Regioni e gli enti locali di trattenere una percentuale della quota recuperata. È quindi, a mio giudizio, estremamente positiva la modifica introdotta con l'approvazione del provvedimento alla Camera dei deputati (articolo 2, comma 1, lettera *d)* e articolo 26, comma 1, che prevede un sistema premiale per le Regioni e per gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto all'elusione fiscale. In conclusione, con l'approvazione definitiva del federalismo fiscale si raggiunge un obiettivo storico per il nostro Paese: una formazione politica come la Lega, assieme ai propri alleati e ai Gruppi parlamentari che hanno dato la propria adesione, ottiene un risultato che è stato perseguito da anni e che rappresenta anche la ragione stessa iniziale della propria esistenza come formazione politica autonoma, legata al territorio. Il federalismo è un'assoluta novità per l'Italia, apre quindi una nuova prospettiva nella coalizione di Governo ed instaura tra PdL e Lega una più stretta collaborazione. Esiste oggi, in altri termini, un'ulteriore opportunità politica e programmatica da parte della maggioranza di Governo e allora forse è possibile avviare un processo storico capace di instaurare in Italia un

a far dimenticare a larghi strati del popolo italiano che avete governato ininterrottamente dal 2001 al 2006, ma io non lo dimentico: quegli anni sono stati persi e, conseguentemente, siamo già in ritardo.

motivo rischiare di fare un lavoro zoppo quando potremmo fare un bel lavoro? Non c'è nessuno qui dentro che pensa che questa sia una cosa intelligente; allora, modifichiamo

agli emendamenti, sono stati presentati anche alcuni ordini del giorno che esprimono la nostra preoccupazione e l'impegno che vorremmo ottenere dal Governo perché sentiamo il grido di dolore proveniente dagli enti locali.

il ministro Tremonti, ma non solo lui, perché, tanto per dire, il ministro Gelmini sta governando la scuola a colpi di circolari facendoci rimpiangere la Falcucci, che almeno le circolari sapeva farle, per non parlare

non vogliamo, tra cinque anni, quando entrerà in vigore il pacchetto completo dei decreti delegati, trovarci stremati e senza risorse. La battaglia che abbiamo fatto fatto (una sorta di filo conduttore) per evitare che attraverso questo strumento si creino i presupposti per uno Stato sociale minimo, almeno per tutta la parte che riguarda il *welfare* locale, è per noi una preoccupazione ancora viva,

*(LNP)*. Signor Presidente, ministro Calderoli, onorevoli colleghi senatori, è per me una grande emozione, anche e soprattutto a livello personale, poter intervenire qui oggi, in quest'Aula, come neoparlamentare ad un anno esatto dall'inizio di questa XVI legislatura,

che annunciava l'affermazione del nostro giornale nel panorama dell'editoria quotidiana sull'intero territorio. Oggi per me, e non solo per me, si corona un altro sogno: quello di poter ringraziare ancora una volta il ministro Umberto Bossi, ideatore di quel grande progetto iniziato 25 anni fa e che si chiama Lega Nord. Oggi raggiungiamo un traguardo importante, quello del federalismo fiscale, che rappresenta però solo una delle tappe per la realizzazione del suo progetto, del progetto di Umberto Bossi, che noi tutti condividiamo e per la cui realizzazione siamo oggi chiamati qui a contribuire. Una realizzazione Una realizzazione che, se pur con la firma chiara e nitida della Lega Nord, vede la condivisione di tutte le forze politiche in Parlamento, è anche merito del grande processo culturale che è stato portato avanti in questi anni, sempre a testa alta, dalla Lega Nord. Si tratta, infatti, di uno dei temi centrali di questa legislatura: il federalismo fiscale attraversa, infatti, tutte le principali politiche pubbliche, da quelle economiche, tributarie, sociali a quelle infrastrutturali, per riassumere in sé i diversi profili, nella scuola, nella pubblica amministrazione, nell'organizzare forme di solidarietà o spazi culturali che condizionano lo stesso modo di essere e di atteggiarsi del sistema integrato Stato, autonomie ed Unione europea. È la prima volta nella storia di questa Repubblica, come ha già sottolineato in quest'Aula del Senato in prima lettura il nostro presidente senatore Bricolo, che una riforma così importante per lo Stato non è stata motivo di contrapposizione politica. Anzi, in Commissione, il testo è stato approvato senza alcun voto contrario. Non era mai successo. Il federalismo fiscale costituisce quindi una tappa determinante di una lunga trasformazione politica ed istituzionale, una trasformazione che la Lega Nord sta «chiamando» da tempo, ma che solo oggi, con il superamento di tanti pregiudizi o chimere da parte di chi nell'attuazione del federalismo vedeva una conseguente distinzione tra Regioni di serie A o di serie B o un eccessivo aumento della spesa e della tassazione a carico dei cittadini; con il superamento, appunto, di questi pregiudizi, siamo finalmente riusciti a portarlo nelle Aule parlamentari per renderlo realtà. Attraverso il federalismo fiscale l'esercizio dei poteri pubblici sarà sempre più vicino ai cittadini, grazie ad un graduale passaggio da una rigida centralizzazione amministrativa alla compiuta valorizzazione e responsabilizzazione del sistema delle autonomie. Perché è proprio grazie al federalismo fiscale che l'imposta si fa più territoriale, più vicina alla gente che non si fida più di chi amministra i suoi soldi dai Palazzi o dalle stanze dei bottoni. La maggioranza dei cittadini ci chiede oggi forme di governo più concrete, più vicine al territorio in cui vivono. Grazie a questo stretto legame che unirà il cittadino alla finanza pubblica ogni cittadino, infatti, saprà come verranno spesi i soldi che paga in imposte e quali saranno le destinazioni delle imposte stesse a favore del proprio territorio. Ecco, quindi, perché parliamo di territorialità dell'imposta che va anche e soprattutto nella direzione di una maggiore responsabilizzazione degli amministratori locali. Un discorso, questo, che posso ben comprendere e condividere come Sindaco di San Genesio ed Uniti, un piccolo Comune alle porte di Pavia, dove fino ad oggi io - come tutti gli altri Sindaci - ho sempre dovuto dipendere, per quello che riguarda per esempio la realizzazione di opere pubbliche o l'erogazione dei servizi, dai trasferimenti dello Stato centrale. Ora, grazie al federalismo fiscale, i sindaci avranno risorse dirette cui attingere e renderanno quindi conto del proprio operato direttamente ai loro cittadini. Il disegno di legge che ci stiamo apprestando ad approvare rappresenta quindi una tappa fondamentale di un complesso processo di transizione del nostro ordinamento verso forme più moderne ed efficienti di esercizio della sovranità popolare, ed è il frutto di un intenso lavoro istruttorio, portato avanti con determinazione e tenacia dal Governo, ed in particolare ricordiamo il grande lavoro del ministro Calderoli, in stretta collaborazione con le autonomie territoriali e perfezionato poi dal Parlamento. Stiamo parlando di un federalismo fiscale equo, intelligente, prudente, trasparente e di orientamento europeo, ma anche solidale e cooperativo, fondato sulla sussidiarietà e la leale collaborazione tra i livelli di governo; diretto a modernizzare l'intero apparato pubblico, responsabilizzando, cosa molto importante, come ho già detto prima, i Governi e le classi dirigenti locali nella cura e nella tutela dei diritti fondamentali e degli interessi collettivi. Con il federalismo fiscale, poi, si applicherà un graduale passaggio dal sistema dei trasferimenti fondato sulla spesa storica, che altro non è se non la sommatoria delle inefficienze a dei costi effettivi, a quello dell'attribuzione di risorse basate sull'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard necessari a garantire sull'intero territorio nazionale il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali degli enti locali. Con il federalismo fiscale le tasse non andranno più tutte allo Stato centrale - lo sappiamo bene - ma si darà finalmente piena autonomia finanziaria ai nostri Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni. Ciò avverrà senza costi aggiuntivi per i cittadini, con la diretta conseguenza di una sostanziale diminuzione del prelievo fiscale: lo Stato chiederà meno tasse. Questo significa che si supererà, per tutti i livelli istituzionali, il criterio della spesa storica, per passare ad un'unità di misura basata appunto sui costi delle prestazioni effettivamente sostenuti a livello territoriale. Altro grande punto di questo disegno di legge concerne i criteri dell'efficienza e dell'efficacia dove i costi reali delle gestioni migliori faranno da riferimento, al fine di costruire un sistema di finanziamento in grado di eliminare le sacche di inefficienza e di promuovere i comportamenti virtuosi, garantendo nel contempo i livelli e la qualità dei servizi resi ai cittadini. Non vorrei sembrare banale, ma vorrei esprimere qui un concetto che credo troverà il riscontro di tutti in quest'Aula: non è giusto che meno si lavora e più si ha diritto di ricevere. Attraverso poi gli indicatori di efficienza e di adeguatezza, volti appunto a garantire obiettivi qualitativi dei servizi regionali e locali, potranno essere strutturati sistemi di riconoscimento per gli enti che assicurano una più elevata qualità dei servizi associata ad un livello di pressione fiscale inferiore alla media, mentre nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e che non adottano le misure correttive necessarie, incluso l'utilizzo dei margini disponibili di incremento del prelievo, è prevista la definizione di un sistema sanzionatorio (perché è giusto che chi sbaglia paghi), giusto che chi sbaglia paghi), che contempla il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali. Non è secondario che il federalismo fiscale venga varato in una situazione finanziaria così preoccupante. Un sistema che parte dal basso, dalla periferia, è sicuramente in grado di meglio competere sul fronte dell'economia. Non solo, ma ricordo, come ha sottolineato nel suo intervento in prima lettura il collega senatore Vaccari, che se tutto il Paese applicasse gli standard e la spesa del Veneto e della Lombardia, già ora avremmo ogni anno circa 3 miliardi di euro di risparmi e di minore spesa a parità di servizi e di qualità, che sarebbero anzi tra i più eccelsi, essendo riconosciuta a livello mondiale la grande validità degli standard di queste Regioni. Concludo con una considerazione finale che reputo essenziale: il federalismo fiscale rappresenta quella scelta politica fondamentale per il reperimento delle risorse finanziarie senza le quali Comuni, Province e Regioni non possono svolgere le funzioni di cui sono titolari.

il provvedimento che ci apprestiamo a varare quest'oggi rappresenta per il nostro Paese una svolta di portata straordinaria. La

che trasforma il sistema politico e istituzionale sulla base di un principio ben definito, quello di responsabilità. Questo perché realizza più democrazia, più controllo diretto da parte dei cittadini, riportando ai livelli di ogni singolo governo, quanto più possibile, la responsabilità della spesa e dell'entrata.

momento si provocò uno scollamento tra il momento della responsabilità verso i cittadini della raccolta fiscale e quello della raccolta di consenso e dell'assenso presso gli stessi attraverso la distribuzione della spesa pubblica.

ma la sua attuazione è stata incompleta soprattutto perché, per lungo tempo, non è stato applicato l'articolo 119 della Costituzione. Se uno dei principali obiettivi della riforma federalista era ed è la valorizzazione del principio di responsabilità, non era sufficiente attribuire alle Regioni maggiore autonomia legislativa e amministrativa; occorreva anche cambiare il sistema di finanza pubblica secondo i principi del federalismo fiscale. solo dando alle Regioni autonomia finanziaria sul versante delle entrate e delle spese, garantendo al tempo stesso il potere tributario sulle basi imponibili agli enti locali ed ancorando il tributo alla territorialità sarà possibile valorizzare il principio di responsabilità. la responsabilità politica indotta dal federalismo fiscale potrà permettere di raggiungere alcuni obiettivi ben definiti: in primo luogo, quello dello sviluppo di politiche realmente rispondenti ai desiderata dei cittadini. Si crea così un meccanismo che potremmo definire di incentivo istituzionale, affinché i governi substatali utilizzino le risorse ottenute con il prelievo fiscale per corrispondere davvero alle aspettative e ai bisogni della cittadinanza. Si crea, inoltre, una sorta di competizione virtuosa tra le Regioni perché gli abitanti di ciascun territorio potranno giudicare comparando i diversi governi regionali, valutando i risultati della propria Regione anche sulla base dei comportamenti tenuti da altre Regioni, ed in questo modo si crea uno stimolo alla diffusione delle pratiche più virtuose. Infine, come conseguenza di quanto detto, ci sarà anche un disincentivo nei confronti delle pratiche amministrative inefficienti e dello sperpero di risorse pubbliche. Se, come detto in precedenza, il principio di responsabilità è elemento centrale di questo provvedimento, lo stesso, in ogni caso, dovrà confrontarsi con un altro principio ugualmente importante per il nostro assetto costituzionale: il principio di uguaglianza dei cittadini, di tutti cittadini, quale che sia il territorio di residenza. Principio che sul piano della struttura federale si traduce nella norma costituzionale secondo la quale in tutto il Paese devono essere garantite entrate sufficienti per finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. La conseguenza sul piano delle tecniche del federalismo fiscale è la necessità di un fondo perequativo destinato ai territori con una minore capacità fiscale per abitante. Il federalismo fiscale si gioca, infatti, nell'equilibrio tra le ragioni dell'autonomia e quelle della solidarietà: solo così potrà servire e valorizzare il principio di responsabilità garantendo al tempo stesso l'unità nazionale. Ed a questo equilibrio si affida il delicato compito di dare una risposta al cruciale quesito di ogni comunità democratica: come garantire l'unità politica nonostante le differenze e, inversamente, come tutelare le differenze nonostante l'unità? Se federalismo e federalismo fiscale, in particolare, servono a raggiungere tali obiettivi, se è nostro dovere dare risposte adeguate al problema dell'equilibrio tra unità e differenza, il disegno del federalismo fiscale deve fornire giuste risposte al malessere del Nord, ma non può dimenticare il Mezzogiorno d'Italia. effettivamente vincere la sfida della competitività in Europa e nel mondo, non può restare con un terzo della propria popolazione e del proprio territorio in uno stato di sviluppo inadeguato, un territorio, il Mezzogiorno, in cui il prodotto *pro capite* è risultato solo poco superiore al 50 per cento del prodotto *pro capite* del Centro-Nord mentre il tasso di disoccupazione è tre volte superiore ed il reddito medio è di gran lunga inferiore. E non voglio in questa sede fare analisi del come e perché si è creato questo squilibrio, non sono questi la sede ed il momento giusti, anche se sono convinto che le radici di queste situazioni risalgano all'Ottocento e in quello che molti storici hanno definito il processo di mala unità. Tornando all'argomento, credo che il federalismo fiscale, se coniugato con principi di responsabilità e solidarietà, possa essere chiave di volta anche per il Sud. Sud. Il federalismo fiscale serve anche al Sud perché responsabilizza la sua classe politica e pone un incentivo all'uso efficiente delle risorse, anche se al tempo stesso è impensabile che da solo il Sud possa farcela da solo a colmare il divario. Per questo è stato quanto mai opportuno introdurre il fondo perequativo e per questo servono gli interventi aggiuntivi previsti dall'articolo 119 della Costituzione secondo cui, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e promuovere la coesione, lo Stato lo Stato stesso finanzia interventi speciali per determinati Comuni, Province, città metropolitane. Altrettanto opportuna allora è la presenza dei due fondi di perequazione in modo che gli enti locali abbiano certezza e contezza delle risorse che arrivano direttamente alle comunità locali. Ed allora la sfida del federalismo fiscale si gioca nell'equilibrio tra le ragioni dell'autonomia e quelle della solidarietà. Occorre dunque essere pienamente consapevoli che soltanto quando sarà stato eliminato il grande divario tra Nord e Sud potremo completare il percorso virtuoso di un federalismo che, pur di valorizzare le specificità e le risorse di ogni singolo territorio, riesca al tempo stesso a garantire l'unità del Paese poiché è in grado di assicurare ad ogni Regione pari condizioni territoriali di sviluppo in termini di servizi. Ma per cogliere questo obiettivo sono necessarie scelte che vadano verso un riequilibrio non solo in chiave economica, ma anche strutturale ed infrastrutturale non è pensabile uno sviluppo senza infrastrutture e una crescita economica senza rapidità nei collegamenti. Anche qui vi è una forbice da dover recuperare se consideriamo, ad esempio, che l'indice sintetico di dotazione di infrastrutture per la mobilità indica per il Mezzogiorno un valore pari a meno della metà di quello del Centro-Nord.

che deve poter contare sulla volontà della politica, sulla semplificazione delle procedure di erogazione delle risorse pubbliche, sull'impegno e la capacità delle Regioni meridionali ad utilizzare i cofinanziamenti comunitari in termini di maggiore tempestività e selezione qualitativa degli interventi, e in chiave microsettoriale ma su grandi e significativi progetti. Saper comporre un quadro organico ed equilibrato: questa è la sfida che la riforma del federalismo fiscale dovrà vincere. Se vincerà questa sfida supererà anche le difficoltà e i rischi di cui parlavo all'inizio. Se vincerà, vincerà l'intero Paese.

dalla Camera, come in fin dei conti ricordato anche dal relatore. La mancata presentazione contestuale della Carta delle autonomie sancisce un federalismo penalizzante, soprattutto per i territori più deboli del Sud d'Italia, perché il federalismo si esaurisce soltanto nell'aspetto fiscale, trascurando l'assetto istituzionale, che invece doveva essere contestuale, o addirittura doveva rappresentare il presupposto del federalismo fiscale. Introduce interventi di privilegio - e, dunque, di disuguaglianza - con l'inserimento, veramente strano ed estraneo alla materia, di Roma Capitale, il trasferimento a titolo gratuito dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato e, soprattutto, la sottrazione allo Stato stesso di importanti competenze. Non parliamo poi dell'introduzione di altre Città metropolitane che non capiamo quali presupposti possano avere per essere considerate tali. Non definisce con chiarezza le funzioni per l'istruzione e, dunque, i relativi capitoli di spesa; esclude il trasporto locale dalla spesa per i livelli essenziali delle prestazioni; non prevede meccanismi adeguati ad evitare il rischio di un aumento della pressione fiscale a carico dei cittadini e delle imprese; non garantisce l'assistenza sociale e sanitaria in maniera omogenea, così come prevede la nostra Costituzione, a tutte le Regioni, in quanto risultano ancora penalizzate Regioni, come quelle del Mezzogiorno d'Italia, nelle quali il numero degli anziani è molto rilevante rispetto al numero degli ospedali, parametro che evidentemente privilegia Regioni nelle quali, invece, il numero degli ospedali è di gran lunga più rilevante. Il Parlamento continua ad essere escluso di fatto dalla cabina di regia di attuazione della riforma ed esiste ancora molta genericità nella definizione dei costi standard da finanziare proprio con questo federalismo fiscale. Non è recepito - e questo è un aspetto che ricordo ancora una volta, ma che probabilmente non interessa granché - il tema della territorialità dell'imposta. Credo che non sia stato affrontato nella maniera più giusta

L'IRPEF deve essere pagata dove viene prodotto il reddito e non dove ha sede legale l'azienda. Penso - lo dico ai miei amici pugliesi - al problema dell'Ilva di Taranto,

lavorando nella città di Taranto e certamente non possiamo essere contenti di qualche posto di lavoro che si traduce più che altro in cassa integrazione piuttosto che in posti di lavoro stabili per la città di Taranto. Non fornisce informazioni ufficiali sui costi, sicché l'applicazione della riforma si potrebbe tradurre in un'inutile moltiplicazione di centri di spesa e di potere con costi aggiuntivi di decine di miliardi di euro.

che il Ministero dell'agricoltura, che è stato cancellato due volte per *referendum*, non soltanto continui ad esistere, senza che siano invece state delegate le funzioni alle Regioni che hanno titolo

Abbiamo ricordato spesso il tema delle responsabilità degli amministratori, cosa giustissima, ma non abbiamo toccato le responsabilità che competono allo Stato nel momento in cui impone con legge il federalismo fiscale, che presuppone una forte organizzazione in termini di uomini e strutture. È disposto lo Stato a trasferire a Regioni ed enti locali uomini e mezzi per controllare e riscuotere i propri tributi? È disposto a formare e ad aggiornare a proprie spese il personale amministrativo preposto agli uffici del fisco? È disposto a creare una magistratura tributaria per garantire al cittadino contribuente di potersi difendere in una posizione di parità dal fisco? Sono tutte domande ad oggi senza risposta, perché, di fronte ad una legge che detta solo principi generali, non si è in grado di fornire dei dati sugli effetti finanziari della riforma, né sul grado di maggiore responsabilizzazione della classe politica e, più in generale, della classe dirigente. Ciò che noi temiamo nel Mezzogiorno d'Italia non è il federalismo in sé, che anzi può essere qualcosa di estremamente positivo, perché incentiva all'assunzione delle responsabilità in un rapporto molto più corretto tra il cittadino e le istituzioni. Quello che temiamo è l'attuale azione di Governo. Per dirla in soldoni, non vorremmo che fra due anni ci dovessimo trovare con i decreti attuativi del federalismo fiscale, con i fondi FAS dirottati altrove e addirittura con i fondi comunitari che dovrebbero essere destinati alle Regioni dell'obiettivo convergenza dirottati nelle Regioni del nel qual caso, a noi rimarrebbe semplicemente il federalismo fiscale, con tutte le sue tasse. In conclusione, su questo disegno di legge c'è da dire una cosa in termini squisitamente politici. C'è veramente da togliersi il cappello di fronte agli amici della Lega

non più relegato soltanto nella macroregione del Nord, ma partito che legittimamente si può estendere su tutto il territorio nazionale, in quanto immagina un'Italia federale. È su questa Italia federale, da costruire realmente nei contenuti, che in futuro si può lavorare. però questo provvedimento non è da me condiviso nei contenuti, anche se con grande attenzione guarderemo ai percorsi che la Lega seguirà nell'assetto di un'Italia federale, che rappresenta il grosso risultato politico che quel partito giustamente può portare a casa.

il federalismo è una riforma che deve realizzare l'uguaglianza vera degli italiani, dal Nord al Sud del Paese. Traguardo ambizioso, che si raggiunge, nel pieno rispetto del nuovo Titolo V della Costituzione varato nel 2001 dal centrosinistra e approvato poi dal *referendum* popolare, inquadrando il federalismo in una cornice fiscale equanime, senza disparità tra le varie aree del Paese. Il che vuol dire attuare un equilibrio tale da scongiurare il rischio che le Regioni a più bassa capacità fiscale abbiano perdite più consistenti. e il PD ha più volte manifestato la propria contrarietà ad un'ipotesi del genere - l'applicazione del Titolo V della Costituzione si configurerebbe come una punizione nei confronti delle comunità residenti nei territori regionali più deboli. invece bisogna tornare alla Costituzione e recuperare il principio di uguaglianza dei cittadini, sancito dall'articolo 3, per garantire la coesione del Paese e rafforzare l'unità nazionale. Ancora, sempre nel quadro dell'attuazione del Titolo V della Parte II della Costituzione, occorre recuperare l'articolo 119, in base al quale «la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante». Il federalismo va inquadrato nell'ottica di una riforma costituzionale complessiva, nella quale venga dato grande rilievo alle autonomie locali, in una logica di perequazione fiscale e tributaria. Bisogna puntare sulla presenza forte dello Stato mediante un rapporto più stretto tra istituzioni centrali e periferiche, assunto che la perequazione finanziaria tra Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni deve necessariamente essere in capo allo Stato per evitare che sul piano dei tributi risultino avvantaggiate le Regioni più forti. Decentrare e trasferire i poteri verso il basso può risultare decisivo per il futuro del Mezzogiorno, con una conseguente maggiore assunzione di responsabilità da parte delle classi dirigenti del Sud. Il federalismo, se ispirato a principi di equità, può contribuire in misura determinante a risollevare le sorti del Sud, evitando che affondi nelle sabbie mobili della criminalità, che ha a disposizione risorse ingenti per controllare l'economia dei territori. Anche per questo, soprattutto in materia fiscale, occorre passare dalla spesa storica alla spesa standard, ma gradualmente e sul piano dei fatti, con un triennio preventivo per recuperare il ritardo del Sud rispetto alle aree più sviluppate del Paese. Destano più di qualche preoccupazione i dati SVIMEZ, che prevedono che con l'attuale disegno di legge del Governo vi sarà uno spostamento di risorse per un miliardo di euro dal Sud al Nord del Paese. Altro che politica per il Mezzogiorno da parte del Governo Berlusconi! Per questo non può non confortarci l'approvazione alla Camera della mozione dell'onorevole Franceschini, che prevede un allentamento del Patto di stabilità interno per consentire agli enti locali di sbloccare fondi disponibili per il pagamento di opere già realizzate, cantierate o programmate. In tal modo, si darà un po' di respiro, soprattutto agli enti locali del Sud, che devono fare i conti con tagli sempre più consistenti. Il Governo a parole celebra le bellezze del Sud e raccoglie consensi nel Mezzogiorno, ma nei fatti sottrae al Sud sempre più risorse, decurtando il Fondo per quasi che il Sud, con le sue enormi potenzialità, solo parzialmente espresse, non fosse parte integrante del sistema Paese. Con questa mentalità il federalismo non ha senso, se non quello, in verità assai poco democratico, di acuire le differenze e allargare le distanze tra aree più efficienti e aree meno efficienti del Paese. Per questo, in una logica di federalismo equo e perequazione tributaria, Regioni e Province a Statuto speciale vanno inserite in un regime ordinario. Infine, la delega dell'attuazione che viene assegnata al Governo ci deve far riflettere, perché far riflettere, perché dovrebbe essere attribuita ad una Commissione interistituzionale (composta da senatori, deputati e rappresentanti di Regioni, Province e Comuni) non essere una delega senza possibilità di controllo preventivo e di verifica costante. In questo modo si realizza il coinvolgimento necessario a rendere il federalismo una riforma del Paese per tutto il Paese,

Con l'approvazione del federalismo fiscale possiamo avere un Paese equo, dando al Mezzogiorno l'opportunità di una straordinaria risorsa, che non è solo per il Mezzogiorno ed il Mediterraneo, ma per l'intero Paese. In un contesto europeo allargato, solo così possiamo affrontare le sfide globali e planetarie che oggi il nostro Paese e l'Europa intera hanno di fronte.

Signor Presidente, signori del Governo, colleghi senatori, l'inizio del percorso parlamentare sul federalismo fiscale è coinciso con i momenti più virulenti della crisi economica e finanziaria che ancora lacera il mondo intero e che, salvo flebili segnali, non intende mostrare ancora segni di inversione di tendenza. Proprio in quei momenti alcuni commentatori delle vicende socio-politiche del Paese levarono le loro voci accusando Governo e maggioranza parlamentare di superficialità: scompaiono i posti di lavoro, dicevano, e il Parlamento si dedica al federalismo fiscale, anziché pensare all'occupazione, alla famiglia, ai nuovi emarginati. Una cultura, questa, che è la medesima che ha condotto il Paese sull'orlo del baratro finanziario negli anni del debito pubblico, del pensiero dell'oggi al di sopra di ogni cosa, dell'insofferenza rispetto a comportamenti virtuosi. Uno dei pericoli più presenti nelle aziende che affrontano un lungo periodo di crisi consiste nella facile e miope soluzione che tende a contrarre le risorse per gli investimenti allo scopo di sostenere le spese correnti. Se il fenomeno si protrae nel tempo l'azienda si emargina dal mercato perdendo competitività in innovazione, tecnologia, qualità, spazi commerciali. L'Italia è un'azienda in crisi perché non ha saputo rinnovare nel tempo il proprio capitale investito, o lo ha fatto solo parzialmente.

Si tratta del sistema nel suo complesso, composto da capitale istituzionale, da legislazione corrente, da organismi pubblici, dalle relazioni economiche e fiscali, dai servizi, dall'economia, dal tessuto sociale, dal contesto ambientale. La legge sul federalismo fiscale, alla quale dovranno seguire Carta delle autonomie e riforma costituzionale dello Stato in senso federale, rappresenta un investimento un investimento ineludibile che, al contrario di quanto sostenuto dalle immote cassandre conservatrici, rimodella i rapporti fiscali tra Stato, autonomie, cittadini secondo il principio della responsabilità. Se il federalismo fiscale fosse stato in vigore all'inizio degli anni Ottanta sicuramente non dovremmo oggi, in questo periodo di crisi, fronteggiare l'emergenza correndo con le mani legate dietro alla schiena, a causa di un debito pubblico che che supera i 1.700 miliardi di euro ed una spesa pubblica che rappresenta circa il cinquanta per cento del PIL. Come tutti gli investimenti, anche il federalismo fiscale non potrà esplicare i propri effetti precipui e specifici che lo contraddistinguono, immediatamente; ma il fatto che sulla qualità del progetto e sugli obiettivi da raggiungere ci sia stata una convergenza parlamentare di amplissima portata, quasi sconosciuta nella storia repubblicana, offre al Paese un segnale importantissimo. Colleghi, abbiamo saputo volare un po' più in alto rispetto alle questioni dei costi della *buvette*, e va dato atto e merito di ciò a tutte le forze politiche che vi hanno contribuito. Che di questo segnale sia innegabilmente promotore ed artefice un movimento politico autonomista e federalista come la Lega Nord, che rappresenta i cittadini di una parte del Paese, sta a significare che quando si fanno delle scelte politiche di grande valore e che danno attuazione alla propria profonda coscienza del bene comune, si guarda al futuro senza alcuna reticenza, senza pensare di essere o non essere masochisti; senza, come dicevo all'inizio, lo sguardo miope sull'oggi. Da domani il Paese, grazie alla legge sul federalismo fiscale, sarà diverso, inizierà un percorso virtuoso, complesso ed articolato, che coinvolgerà la responsabilità degli amministratori locali, che aggredirà la mole della spesa pubblica, che guiderà cittadini ed imprese verso un ruolo attivo e attento nei confronti della pubblica amministrazione. È quello che ci hanno chiesto i cittadini col voto di un anno fa e che chiedono a piena voce ancor più oggi; più è quello che chiedono i cittadini del futuro, magari non ancora nati, o i bambini o i giovanissimi, tutti quelli che saranno costretti a portare sulle proprie spalle l'inefficienza del passato se non avremo la forza e il coraggio di completare in tempi accettabili il percorso iniziato nel 2001 con la riforma del Titolo V, che continua oggi con il federalismo fiscale, che deve proseguire incidendo profondamente nell'architettura delle istituzioni.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione ha generato un ampio e costruttivo dibattito in Parlamento e nel Paese, anche grazie al coinvolgimento dell'opposizione. Il tenore e la portata di tale provvedimento ha infatti imposto una riflessione politica e culturale, che va dalla revisione della contabilità dello Stato alle riforma del sistema degli enti locali, dalla ridefinizione del concetto di solidarietà tra i territori all'introduzione del tema di una riforma istituzionale e costituzionale. Con questo atto il Governo ha deciso di affrontare la pericolosa inerzia del *trend* del deficit pubblico e dell'evasione fiscale, varando una riforma che, a partire dagli aspetti fiscali e amministrativi, ha l'ambizione di porre le premesse di una compiuta trasformazione in senso federale del sistema istituzionale italiano. Il federalismo fiscale si propone perciò quale primo tassello di una nuova fase costituente, che potrà svilupparsi in modo analogo a quanto avvenuto sul piano delle istituzioni comunitarie, dove, partendo da elementi economici e finanziari come l'introduzione dei parametri di Maastricht prima e l'unità monetaria poi, ci si è posti l'obiettivo di una vera e propria Costituzione capace di rispecchiare l'evoluzione avvenuta nella politica e nel costume dei popoli europei. Una nuova fase costituente del resto ineludibile, perché conferendo a Regioni ed enti locali una rafforzata soggettività attraverso una più ampia capacità impositiva, il delicato sistema di pesi e contrappesi disegnato dalla Carta del 1948 andrà inevitabilmente erodendosi, perdendo vieppiù efficacia. L'intervento sulla Costituzione dovrà pertanto essere teso ad evitare la frammentazione diretta e indiretta dei centri decisionali, eventualità questa che comporterebbe ricadute nefaste sulla sintesi amministrativa necessaria ad un'adeguata capacità di Governo. Il federalismo fiscale presuppone, insomma, l'avvio di una nuova fase costituente, poiché semplificando il patto fiscale tra cittadini e livelli di Governo territoriale è impensabile mantenere un impianto costituzionale che contempla dalle 23 alle 29 materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni. In questo senso, lasciare inalterato il Titolo V vanificherebbe infatti i caratteri di effettività e responsabilità introdotti in maniera esplicita dalla presente legge delega. Siamo perciò di fronte ad una vera e propria rivoluzione che trasformerà un sistema centralizzato, e sostanzialmente irresponsabile nel suo fondarsi unicamente sulla spesa storica, in un sistema articolato, modellato dal criterio di costi e fabbisogni standard, i cui meccanismi premiali per Regioni ed enti locali virtuosi saranno oggetto di positiva competizione tra territori. Bisognerà tendere ad un ottimo per garantire, non solo sulla carta, una sorta di tetto fiscale tra tributi locali e nazionali, al fine di non oltrepassare un dato limite (che potrebbe essere, ad esempio, quello del 40 per cento), oltre il quale il Paese sarebbe condannato alla crescita zero. Allo stesso modo, sarà opportuno stabilire con precisione competenze in materia di interesse locale, provinciale, regionale e nazionale e vigilare in sede di Commissione bicamerale affinché tale ripartizione sia rigorosa, onde scongiurare quella moltiplicazione di fattori di spesa pubblica che finirebbe per aggirare i parametri imposti dal concetto di costi standard. È una sfida, colleghi, difficile e pur necessaria, ma viste le innovazioni introdotte durante il passaggio parlamentare del testo in esame possiamo dirci ottimisti circa un equilibrato e sostenibile processo transitorio. Da senatore toscano vorrei poi testimoniare la mia soddisfazione per l'inserimento di Firenze tra le aree metropolitane previste da questa legge. L'introduzione di un nuovo livello di governo, sostitutivo delle Province come appunto l'area metropolitana, se non significherà automaticamente più risorse per il territorio fiorentino si tradurrà comunque, se ben recepita, in strumenti e procedure più efficaci per affrontare quelle sfide dello sviluppo, non sempre colte dalla classe amministrativa locale. Penso in particolare al nodo delle infrastrutture di comunicazione e di servizio, che strozzano lo sviluppo urbano ed economico della mia città. Tuttavia a Firenze, ministro Calderoli, non basta un'area metropolitana: lo dico qui, in sede di approvazione di un testo di legge che configura obiettividi perequazione e solidarietà e che formalizza la legge per Roma Capitale. Dopo i codici speciali per Roma e Venezia, l'implementazione della città metropolitana dovrà rappresentare il punto di partenza per arrivare ad uno statuto speciale di Firenze. Se dal punto di vista perequativo, il capoluogo toscano dà oggi allo Stato più della somma dei trasferimenti ricevuti, non si può continuare ad ignorare le speciali esigenze di una città di 300.000 abitanti, che si trova a ricevere ogni anno oltre 7 milioni di turisti. Per questo motivo ritengo opportuno prevedere un apposito progetto di legge dedicato a Firenze, organico e coerente, certo, con i principi del federalismo fiscale, ma capace tuttavia di affermare la specialità di questa città italiana che tra tante difficoltà ospita e custodisce circa un terzo dei tesori d'arte del mondo. Vorrei, infine, concludere con una citazione dello storico americano Clinton Rossiter, che, a proposito dei *Federalist Papers*, scrisse: «Non c'è felicità senza libertà, non c'è libertà senza autogoverno, non c'è autogoverno senza costituzionalismo, non c'è costituzionalismo senza senso morale». Ebbene, credo che il percorso avviato oggi con una legge di riforma tributaria e amministrativa sia in grado di rinnovare non solo il sistema dei rapporti tra Stato e territori in maniera responsabile e solidale, ma anche lo spirito civico ed il senso morale del nostro Paese.

con la terza lettura del disegno di legge delega c'è la necessità, a partire da oggi, di evitare alcuni luoghi comuni per i quali il federalismo, di per sé e in quanto tale, debba essere considerato un punto essenziale obbligato per il riassetto istituzionale dell'Italia o una conquista per i governi locali che vengono chiamati a nuove funzioni. necessario partire da un punto semplice, che è anche il dato politico alla base di questo disegno di legge: tutto dipenderà da come la normativa delegata disciplinerà in dettaglio le misure applicative e insieme ad esse quelle di controllo e quelle sanzionatorie. Siamo d'accordo che un aspetto positivo del disegno di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione consiste nell'introdurre un sistema di responsabilizzazione delle Regioni e degli enti locali; non può funzionare bene un sistema nel quale, da un lato, c'è una diversità di soggetti interessati alla spesa e non corresponsabili delle entrate e, dall'altro, un solo soggetto, il Governo nazionale, tenuto a garantire l'equilibrio del bilancio complessivo. In questo contesto di deresponsabilizzazione che, diciamola tutta, è stato voluto e tollerato da un'intera classe politica degli ultimi decenni, ben venga allora un sistema nel quale chi propone una spesa debba indicare anche le entrate, affermando il principio della corrispondenza tra compiti da assolvere e risorse disponibili.

la spesa *pro capite* delle Regioni meridionali è inferiore di diversi punti rispetto a quella delle Regioni settentrionali, mentre la pressione tributaria riferita a tributi erariali e addizionali regionali risulta in diverse Regioni del Sud pari o superiore In parole semplici: al Sud si spende meno e si tassa ugualmente. Riteniamo, signor Ministro, al di là dei toni solenni, che sarà possibile giudicare compiutamente questa riforma solo quando se ne vedranno i risultati concreti; solo quando potremo constatare se saranno evitati i rischi, paventati da molti, di trovarci con più tasse, più spesa, più debito pubblico, più conflitti dentro la pubblica amministrazione. Il parametro essenziale per noi dell'Italia dei Valori, con il quale valuteremo questo disegno di legge, sarà soltanto quello del pragmatismo, cioè la verifica costante e continua se esso semplicemente funziona. Lo abbiamo dimostrato con il nostro precedente voto di astensione al Senato e favorevole alla Camera, perché è evidente che la convergenza - e lo dico al ministro Calderoli al quale ci lega un rapporto di stima e simpatia - si ha quando si è d'accordo sul merito, senza confondere ruoli e conservando inalterate le distinzioni tra maggioranza e opposizione. Questo, tra l'altro, vale anche per il contrario: chi dissente - e noi dell'Italia dei Valori dissentiamo spesso non si oppone, come si vuole far credere, al sistema, bensì ad un singolo provvedimento, ad un singolo disegno di legge, ad una singola riforma. Occorrerà da parte di tutti i colleghi pragmatismo, perché il disegno di legge sul federalismo ha un impianto estremamente complesso. Lo ha più volte ricordato lo stesso Ministro dell'economia: 12 tributi, 5 soggetti della riscossione, 2 fondi di sussidiarietà, 11 princìpi e criteri generali, 8 tipi di procedure attuative, varie commissioni e livelli decisionali. Pragmatismo, perché non c'è dubbio che per l'introduzione e l'attuazione del federalismo fiscale questo sia, se non il momento peggiore, certamente quello più delicato per le conseguenze ancora non prevedibili e di lungo termine della crisi economica. Ci saremmo aspettati che il Governo fosse consapevole che prima della sperimentazione di ampie convergenze sul federalismo fiscale sarebbe stato utile per tutti convergere sull'analisi della crisi e sulle risposte da dare con le decisioni che sono nelle facoltà del Governo. Proprio ora che lo stesso Governo è stato chiamato a rivedere radicalmente le previsioni che ha comunicato alla Commissione europea ai fini del Patto di stabilità, come si è visto nella Nota informativa 2009-2011 trasmessa a febbraio alle Camere, che ha rivisto in senso peggiorativo la percentuale di crescita del PIL nel 2009 e di seguito le stime del deficit e del debito pubblico. Non c'è bisogno qui di ricordare che uno dei pochi studi in materia di costi di un sistema federale fu fatto proprio durante uno dei Governi Berlusconi, e parla di 100 miliardi di euro di allora. Restiamo però ai dati di oggi sulle spese di funzionamento della messa a regime del sistema federale: tenendo fermi da un lato il parametro dell'invarianza fiscale e dall'altro gli indicatori sulle prestazioni, le Regioni potrebbero essere chiamate, dopo il periodo di transizione, a tagli tra gli 11 e i 16 miliardi, con effetti simili anche per Province e Comuni. Nel corso dell'*iter* legislativo noi dell'Italia dei Valori abbiamo chiesto correzioni e soprattutto chiarimenti. Non ci sono ancora del tutto chiare le conseguenze che determineranno sul piano economico e sociale due delle parole chiave della riforma, costi standard e perequazione, che al momento appaiono due tecnicismi dietro cui si possono nascondere diverse insidie. Il finanziamento degli enti locali avverrà attraverso il costo standard che paga solo i servizi, mentre quello storico premiava spesso le inefficienze; ma ben difficilmente il costo standard potrà, per i dati necessari a costruirlo nel tempo, aiutare da solo il problema della spesa pubblica, ossia gli sprechi e le inefficienze. modo, la perequazione nasconde i dubbi di molti rispetto ad un'equa redistribuzione delle risorse nei diversi territori del nostro Paese, perché la perequazione, quantunque perfettibile, non può essere volta a realizzare parità di trattamento dei cittadini delle diverse realtà territoriali, in quanto l'ordinamento autonomistico è per sua natura diversificato. Con i decreti di attuazione poi si dovrà fissare con precisione entità e qualità dei tributi da assegnare a Comuni, Province e Regioni; non ci si può limitare soltanto a compartecipazione al gettito dei tributi erariali, perché di fatto si favorirebbe il ripristino della finanza derivata e il ritorno della spesa storica. Il nostro pragmatismo ci porta quindi a considerare che il disegno di legge all'esame è per il momento un modello teorico condivisibile, fatto di ipotesi, di principi, di combinazioni tributarie, finora senza cifre né percentuali. le questioni che riteniamo essere ancora aperte sono di carattere formale e sostanziale: tra le prime la più importante è quella relativa agli spazi che il Governo darà nei fatti ai poteri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo, prevista dall'articolo 3. Infatti, se è vero che il concorso del Parlamento nell'emanazione di una legge delega si limita essenzialmente al varo della legge delegante e che con i decreti delegati, propri del Governo, il Parlamento non può recuperare ciò che ha concesso nella delega, deve essere altrettanto chiaro che a questa Commissione vanno di fatto riconosciute ed assegnate funzioni vere e reali di compartecipazione alle scelte e non soltanto un ruolo consultivo. Sui punti sostanziali è necessario resti fermo l'impegno che l'inizio dell'attuazione della riforma federale vada di pari passo a quella della Carta delle autonomie locali, nel cui ambito devono essere riportati gli articolati con contenuto ordinamentale, in modo che il federalismo sia una parte di un disegno più ampio di riforma delle istituzioni. Da parte nostra, signori rappresentanti del Governo, è legittimo che restino alcune perplessità, perché vi è un problema di fondo che non va sottovalutato e che sta nella contraddizione tra i programmi federalisti del Governo e la logica centralista di molte scelte politiche fatte dalla maggioranza. Al riguardo l'insufficiente compensazione del minor gettito ICI ai Comuni; il blocco dell'autonomia impositiva per gli enti locali; i tagli ai trasferimenti erariali; una manovra finanziaria restrittiva, tanto che l'ANCI ha lanciato l'allarme che otto Comuni su dieci in Italia rischiano di non rispettare il Patto di stabilità interno nel 2009; i famosi contestati trattamenti di favore per alcune realtà amiche, tra cui i fondi straordinari per Catania e Roma e l'esenzione di quest'ultima dal Patto di stabilità. Sono tutte misure che rappresentano veri e propri strappi, che tolgono credibilità alla reale volontà della maggioranza di fare del federalismo fiscale qualcosa di più di un semplice manifesto elettorale per i prossimi appuntamenti. Riteniamo

l'autonomia locale, in particolare dei Comuni, in un quadro di accresciuta responsabilità. Da questo punto di vista - e solo da questo - esprimeremo le nostre valutazioni sulle azioni future del Governo.

intervenendo il 20 gennaio scorso in occasione della discussione su questo stesso disegno di legge delega in materia di federalismo fiscale, ebbi a dire che esso rappresenta un

Ritengo che la presente versione meriti un credito particolare in tema di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, assistenziali e scolastiche. Ciò consente di poter affermare che in tutto il Paese resterà correttamente garantita l'eguaglianza nella fruizione di tutti i diritti esigibili in forza del novellato testo dell'articolo 117 della Costituzione. L'*iter* parlamentare e le istanze istituzionali recepite costituiscono la prova dell'archiviazione di quelle logiche intese ad ingigantire le differenze e le diversità etnico-territoriali, in perenne e costante violazione dell'unità nazionale stabilita dai precetti costituzionali. Mi pare che, senza la pretesa di essere un costituzionalista (perché in effetti nella legge che oggi verrà licenziata sia stato espressamente assicurato un giusto rilievo alle conclusioni cui era pervenuta la Consulta in tema di applicazione concreta dell'articolo 119 della Costituzione. Si è evitato, cioè, di contravvenire alle indicazioni in tema di riparto delle competenze e si è accolta la linea costituzionalistica intesa a tracciare le caratteristiche di un sistema di finanziamento imperniato sul ruolo perequativo di tipo verticale a cui viene chiamato lo Stato. Si attenuano così le differenze territoriali, mediante l'attribuzione di una maggiore disponibilità di dotazioni finanziarie Il lavoro che abbiamo svolto qui in Senato, in prima lettura, ha prodotto i suoi effetti anche nelle fasi successive, sino a stimolare le consistenti modifiche emendative intervenute alla Camera dei deputati. I colleghi deputati hanno accresciuto l'autonomia impositiva delle Regioni e hanno modificato il finanziamento delle funzioni non essenziali e amministrative. Voglio sottolineare in modo speciale le norme che introducono l'opportunità di prevedere - in sede di decreti legislativi -adeguate forme premiali per quegli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di contrasto dell'evasione fiscale. Ritengo positivo, poi, l'aver attribuito significativi poteri alla Commissione bicamerale competente ad esaminare preventivamente i successivi decreti delegati attuativi

in stretta simbiosi con i costi standard, costituiranno gli elementi di base sui quali calcolare l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, sociali e dell'istruzione. La perequazione esclusivamente verticale avrà come conseguenza di gravare sulla fiscalità generale. In tal modo la sussidiarietà fiscale diviene lo strumento per far emergere le caratteristiche territoriali produttive e instaurerà la cosiddetta manovrabilità fiscale, quale elemento di flessibilità del prelievo tributario correlato al programma complessivo di sviluppo economico della comunità locale interessata. Gli ingenti deficit regionali, che allungano la propria ombra anche su questa nuova legislazione, non si potranno più impunemente produrre perché i cittadini male amministrati se ne accorgerebbero ben presto, essendo chiamati al loro livellamento. La scelta di un federalismo solidale e compatibile, tuttavia, mette il Paese al riparo dai guasti di un federalismo esasperato, perché è finalizzata a ricercare

Tuttavia cambieranno molte cose, alcune già visibili nell'immediato. Per esempio, non esisteranno più i trasferimenti di risorse statali verso le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni, fatto salvo quanto previsto dalle norme transitorie. Né esisterà più il concetto di spesa storica, sostituito da quello del costo standard. Rispetto, poi, alla critica più volte sentita sull'indeterminatezza dei costi, basterebbe richiamare l'intervento del 21 gennaio scorso del ministro Tremonti, quando descrisse il nuovo federalismo come un sistema olistico, complesso come quello del corpo umano. Tuttavia, vorrei anche osservare che l'importanza storica della svolta federalista per il nostro Paese assume le caratteristiche di una scelta profondamente politica. Il federalismo fiscale, per tutti i partiti, è un atto obbligato di rispetto della volontà popolare, nonché condizione ineludibile per rilanciare sul piano dell'efficienza amministrativa molti enti locali e Regioni, rispettandone le singole identità. È una sfida da vincere, senza cedere alle sclerosi ideologiche, con possibilità di correzioni che potranno essere necessarie anche nel lungo periodo. Abbiamo scelto non a caso un federalismo solidale, per rendere tutta l'Italia più moderna, più unita, più europea. *(Applausi del

oggi con l'approvazione del disegno di legge in esame si chiude un'epoca, si chiude una fase di centralismo ed assistenzialismo che ha caratterizzato parecchi decenni della vita del nostro Paese. A partire dagli anni '90 si è avviato un ampio processo di riforma istituzionale volto alla realizzazione di uno Stato federale. Questa spinta al cambiamento era dettata soprattutto dalle esigenze della nostra gente,

purtroppo, però, non si è affrontato adeguatamente il tema del federalismo fiscale. Sul nostro Paese ancora oggi grava il peso del notevole ritardo nell'attuazione delle riforme federali, ritardo che ha portato inevitabili ricadute sulla capacità di spesa delle Regioni e degli enti locali. La mancata attuazione del federalismo fiscale ha di fatto prodotto una situazione di stallo, dovuta soprattutto all'incertezza nell'attribuzione agli enti delle risorse ed alla presenza di un sistema regionale di redistribuzione delle risorse fortemente sperequato, basato sostanzialmente sulla spesa storica e non sulla virtuosità amministrativa. Ciò non ha favorito la responsabilizzazione dei governi locali e l'autonomia degli enti periferici: si è finito per premiare chi più sprecava, mentre si penalizzava chi era efficiente. situazione ha creato un debito pubblico elevato e che - tanto meno oggi, con la crisi economica in atto - non è più sostenibile. È ora di cambiare, bisogna premiare chi fa bene e punire chi sperpera. Questo provvedimento va finalmente in tale direzione, prevedendo che si superi l'attuale sistema basato sulla finanza derivata, ispirato al criterio della spesa storica, per arrivare ad avere invece un sistema pubblico che sia efficace ed efficiente. Importante è anche la previsione che vengano premiati quegli enti che ottengono risultati positivi in termini di lotta all'evasione e all'elusione fiscale, creando un collegamento diretto tra reperimento delle risorse pubbliche e gestione della spesa. Si rafforza sempre più sia il controllo degli enti sui contribuenti, sia il legame tra gli amministratori e i cittadini, che sono in grado di valutare meglio

responsabilizzati, dovranno necessariamente essere più accorti nella gestione della finanza pubblica. Purtroppo finora si è assistito solo ad una realtà in cui non si premiava chi lo meritava: lo meritava: le Regioni virtuose, ad esempio, si trovano costrette ancora oggi a dover rispettare vincoli rigorosi del Patto di stabilità e a finanziare ingenti flussi perequativi verso altre Regioni. Ma con questo provvedimento la situazione migliorerà. Il disegno di legge che approveremo prevede, infatti, un nuovo sistema di perequazione: un sistema alla tedesca, con riduzione delle differenze tra i territori, ma senza alterarne l'ordine nella graduatoria delle capacità fiscali fra prima e dopo la perequazione, limitandosi a ridurre i differenziali di risorse tra le diverse aree. Sono convinta che per favorire lo sviluppo di tutto il nostro Paese sia necessaria una solidarietà che superi la mera logica dell'assistenzialismo e che responsabilizzi i singoli amministratori. A solo un anno dall'inizio della legislatura questo disegno di legge dà attuazione all'articolo 119 della Costituzione e si ispira ad un principio solidaristico, volto alla promozione della crescita e dello sviluppo delle singole realtà territoriali. L'attuazione del federalismo fiscale è una riforma fondamentale per il Paese, condivisa al di là delle diverse posizioni politiche e chiesta a gran voce dalla nostra gente. Personalmente sono particolarmente soddisfatta di come si è svolto il confronto ed il dialogo tra maggioranza e opposizione, a dimostrazione che quando si collabora si possono ottenere importanti risultati. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto a questo progetto e che hanno dimostrato che con il dialogo si possono fare le riforme e i cambiamenti di cui tutti abbiamo bisogno. Signor ministro Calderoli, la nostra gente vuole le riforme. Noi le abbiamo inserite nel nostro programma elettorale e le stiamo realizzando senza divisioni. Soprattutto continueremo a farle per il bene del nostro Paese, facendo seguire alle parole anche i fatti. Dopo un lungo percorso di battaglie della Lega Nord Padania siamo finalmente giunti al traguardo: il federalismo fiscale sarà presto una realtà.

Un lavoro che è partito dalla presentazione di un nostro disegno di legge e che ha visto apporti significativi, alcuni dei quali vorrei citare. Innanzi tutto, l'aver lavorato sull'obiettivo per la convergenza per quanto riguarda i servizi è una delle misure che favorisce il Mezzogiorno del Paese. il coordinamento della finanza pubblica, che allinea finalmente la finanza pubblica tra enti locali, Regioni e Stato. Vi è, inoltre, il ruolo che abbiamo rivendicato della Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, affinché il Parlamento monitori tutto il corso dei decreti legislativi attuativi. Il gettito della riserva di aliquota alla compartecipazione dei tributi erariali, con la priorità stabilita sull'imposta dell'IVA, è un'altra misura che favorisce o può favorire i territori a minore capacità fiscale. Abbiamo chiarito, inoltre, che la fiscalità di sviluppo, così come l'articolo 21 per quanto riguarda le nuove imprese, sia riservata alle aree sottoutilizzate. Abbiamo salvaguardato, infine, i fondi perequativi già destinati alla legge n. 549 del 1995. Abbiamo approvato alla Camera un nostro emendamento, suggerito anche dal lavoro svolto dalla SVIMEZ, che prevede interventi organici, piani mirati e finalizzati di tipo pluriennale per il Mezzogiorno. Infine, ma non per ultimo, anzi per primo, nell'articolo 1 tra gli obiettivi della legge è dichiarato che uno degli obiettivi è quello del superamento del dualismo economico del Paese. Non mi sembra una cosa di poco conto, ma di sostanza. Il Parlamento parla attraverso una legge al Paese, parla delle sue disuguaglianze, ma anche delle sue opportunità. Apre un canale di lavoro, un percorso da attivare proprio attraverso il pieno utilizzo di tutti - sottolineo di tutti - i commi dell'articolo 119. Il Partito Democratico parla a un sistema Paese, ad una sinergia possibile tra Nord e Sud, senza la quale non sarà possibile né superare la crisi economica, né affrontare il vero sviluppo del Paese nella competizione globale, meno il tema delle riforme, se crediamo a queste come un processo sostanziale di innalzamento dei livelli civili, funzionali ed amministrativi di tutto il Paese. È una sfida di modernità che le classi dirigenti del Mezzogiorno possono raccogliere, devono raccogliere per quanto riguarda la responsabilità, la trasparenza, l'uso delle risorse, la qualità della spesa e l'efficienza dei servizi. È una sfida che tutto il Paese deve raccogliere e che questo Governo dovrebbe praticare, affinché i diritti di tutti i cittadini siano uguali dovunque essi nascano. Non quindi una legge per alimentare egoismi territoriali, non per scavare sulle disuguaglianze e nemmeno per lasciare tutto così com'è. Ma la riforma suscita ancora molte preoccupazioni in tanti commentatori, in tante parti del Paese, in particolare nel Mezzogiorno, nelle aree a minore capacità fiscale. Eppure il Sud avrebbe potenzialmente da guadagnare in un processo di riforma che accompagni verso la responsabilità, verso livelli essenziali di prestazioni e di servizi che siano tenuti allo standard dei costi e dell'efficienza rispetto alle altre Regioni e rispetto all'Europa. E allora perché ancora queste perplessità? Perché lavorare per questi obiettivi significa, appunto, investire sul sistema Paese; significa tener conto già da oggi delle disuguaglianze, delle diseconomie, e lavorare per attenuarle. Ma quali politiche strutturali sono state perseguite da questo Governo per il Mezzogiorno? Quale uso scellerato è stato fatto dell'unica risorsa disponibile, qual era quella dei fondi FAS, nell'ambito di una crisi economica che ancor più rischia di penalizzare certe Regioni? certe Regioni? È questo che manca. Manca un'affidabilità della politica verso le aree del Mezzogiorno. Manca un'affidabilità di questo Governo verso il Mezzogiorno. È su questo punto che incalzeremo e continueremo la nostra battaglia.

Se non si affronta il tema delle funzioni, della sussidiarietà, se non si eliminano sprechi, duplicazioni, centri di costo e di potere - e sottolineo, al centro come in periferia - se non si tagliano e non si disboscano questi livelli, la riforma rischia di essere vacua, inutile e dannosa. È stato sottolineato anche in qualche intervento dei colleghi della maggioranza con riferimento al Mezzogiorno. È una riforma nella quale il PD si impegnerà affinché l'articolo 118, la Carta delle autonomie, la riforma dei livelli istituzionali e una politica di rigore e strutturale verso il Mezzogiorno risultino fondamentali per completare, anche e non solo attraverso questo passaggio, un quadro di riforme istituzionali senza il quale nemmeno questa riforma sarà credibile. È con queste perplessità,

ora che il Governo, rinviando il tema del federalismo istituzionale e l'introduzione di una forma di governo di tipo presidenziale, ha deciso di mettere in cantiere il federalismo fiscale con una legge delega, avverto il bisogno di dire parole chiare su una riforma che, se nell'immediato riguarda l'aspetto finanziario, costituisce in realtà l'ultimo anello di una catena, il Titolo V della Costituzione, non a caso fortemente voluto dalla sinistra. Il federalismo di cui si tratta, infatti, costituisce secondo la mia lettura non solo una semplice novità di natura fiscale, ma l'ultimo passo di un radicale cambiamento che, se non accompagnato da altre riforme di struttura, alla fine giova fondamentalmente al sistema di governo locale della sinistra, che dinanzi alle possibili conseguenze delle grandi trasformazioni istituzionali portate dal consolidarsi di una cultura della democrazia governante, ha pensato bene di metterlo in sicurezza con opportune riforme di struttura e costituzionali. È bene mettere subito le cose in chiaro: non ho alcuna obiezione dì principio sul federalismo come attuazione del principio di sussidiarietà, un principio che peraltro risale alla dottrina sociale della Chiesa, al riconoscimento dei corpi intermedi e all'importanza del procedere dal basso, dai singoli e dalle microcomunità. La mia obiezione riguarda la procedura e la convinzione che rappresenta un errore la decisione di non mettere mano contestualmente - dunque accanto, anche se separatamente sia alle correzioni condivise del Titolo V, sia all'attuazione del federalismo fiscale, sia all'introduzione di riforme sulla forma di governo. Perché la penso così? Perché sostengo che è preoccupante una riforma solitaria sul federalismo fiscale? Perché tutto il dibattito sul cosiddetto progetto di Lorenzago e sul *referendum* che ne è conseguito ha messo in evidenza che la riforma attuata del Titolo V ha di fatto scardinato l'assetto costituzionale dalla Costituzione del 1948. Nello stesso progetto di Lorenzago, affrontandosi il problema del federalismo fiscale, con una norma specifica è stata rinviata la sua realizzazione a tre anni dopo l'entrata in vigore della riforma. Lo stesso Bossi dichiarò, il 23 agosto del 2003, intervistato dal «Corriere della Sera» sul punto, che un federalismo fiscale attuato subito, senza una riforma preventiva e organica della Parte II della Costituzione, poteva diventare una porta aperta verso la secessione. Perché manifesto queste perplessità? Perché anche la sinistra, almeno a parole, per esempio con Bassanini, aveva denunciato le distorsioni del Titolo V. Nel libro «Salviamo la Costituzione italiana», di Dino Messina, così afferma Bassanini: «Bisogna ammettere che nel definire le competenze legislative concorrenti, dove il Parlamento fissa i princìpi fondamentali e le Regioni legiferano, agli autori della riforma del Titolo V è scappata la mano. È chiaro che materie come grandi infrastrutture, produzione, trasporti, distribuzione nazionale dell'energia e ordinamento delle comunicazioni

«A mio avviso, alla riforma del Titolo V manca un altro elemento fondamentale comune a tutti gli Stati federali: la cosiddetta clausola di supremazia, la norma di principio per cui il Parlamento nazionale può sempre intervenire in qualunque materia di competenza delle Regioni qualora ciò sia richiesto da una serie di ragioni». Ancora. Se così è, è, se il Titolo V andava aggiustato, migliorato, corretto nella disarticolazione della Carta del 1948, come mai la sinistra in questo contesto non parla più di ritoccare e rimettere a posto il Titolo V?

«Si tratta di un peccato gravissimo della sinistra che, per guadagnare qualche voto presso la Lega e cercare di vincere le elezioni politiche del 2001, si lanciò in una riforma federale della quale il nostro Paese non ha alcuna esperienza e di cui non esiste alcun precedente, perché i Paesi federali funzionano in quanto nascono federali». Ebbene, non sono d'accordo con Sartori su questa tesi:

perché - sono convinto di questo dato - la sinistra è stata sempre tarata sulla presunzione politica di una superiorità soprattutto sul tema costituzionale, tanto da pensarsi come partito egemone. La sinistra, infatti, ha lavorato - eccome! - da tempo per realizzare la riforma che poi ha introdotto nel 2001 nella nostra Costituzione. Voglio citare tre esempi di carattere storico. Il primo mi riguarda personalmente. Sono stato eletto deputato nel 1987 e nominato membro della Commissione parlamentare per le questioni regionali presieduta

di proposte legislative della Lega in questo senso) si parlò in maniera esplicita esattamente delle riforme che nel 2001 sono state introdotte nel Titolo V, in particolare

la Lega non aveva su questo tema proposte specifiche, perché era ancorata a tematiche che rasentavano la secessione, come sappiamo. Ebbene, negli atti di quella Commissione si troveranno tutte le proposte che riguardano la cosiddetta *devolution*. Addirittura anche dal punto di vista terminologico, proprio nella relazione che riguarda una di quelle proposte, si fa riferimento alla necessità di «rivedere radicalmente i poteri dello Stato e di dislocare attraverso la devoluzione di competenze alle Regioni (...)». Per non parlare delle proposte specifiche di dettaglio, che riguardano l'atto finale della Commissione Iotti, laddove si parla della modifica dell'articolo 70 della Costituzione, introducendo la sovranità duale tra Stato e Regioni, e dell'articolo 117, introducendo la competenza di carattere generale delle Regioni rispetto a quella tassativa e specifica dello Stato (appunto, il cosiddetto rovesciamento dell'articolo 117). Ecco perché sono convinto che la sinistra più lungimirante, consapevole di uno scenario nazionale caratterizzato, a causa di alcune trasformazioni che già si vedevano all'orizzonte, da un forte desiderio di democrazia governante che poteva di fatto incidere anche nel governo locale, alla fine si è adoperata per introdurre al momento opportuno un federalismo per cessione di poteri e fiscale, che di fatto - è questa la mia tesi - realizza due modelli socio-politico-istituzionali in grado di vivere autonomamente. Per cogliere il senso di ciò che sostengo, non bisogna mai dimenticare che la sinistra post 1948, non potendo entrare per ragioni internazionali nel Governo del Paese, ha fatto dell'amministrazione locale la ragione della propria sopravvivenza, inventandosi il modello tosco‑emiliano come termine di paragone con il Governo statale. Il '68 ha fatto il resto. La sinistra infatti, sfruttandone l'onda, ha premuto per l'attuazione delle Regioni e per l'adozione di una serie di provvedimenti legislativi che - attraverso la costituzione di enti, sottoenti, strutture collaterali, consigli di istituto, comitati di gestione e di quartiere, agenzie, comunità, consorzi, rappresentanti sindacali hanno determinato con un effetto domino la nascita di un sottosistema politico-amministrativo in concorrenza e potenzialmente in conflitto con quello disegnato nella Costituzione. Ecco perché, secondo me, la sinistra ha fatto saltare l'equilibrio costituzionale della Carta del 1948. E l'ha fatto saltare con alcuni passaggi molto semplici. Innanzitutto facendo saltare la sovranità del popolo, che si esercita nella Costituzione del 1948, attraverso l'articolo 70, con la potestà legislativa del Parlamento. Amici della sinistra che non seguite questi temi, sia ben chiaro che con la riforma del 2001 non è più così.

che prima venisse lo Stato e poi le autonomie, mentre in quello del 2001 emerge l'idea per cui lo Stato è una istituzione della Repubblica, a pari dignità con Comuni, Province, aree metropolitane e Regioni». E quando si parla di senso dello Stato o di Capo dello Stato chissà a cosa ci si riferisce. Questa riforma il centrosinistra l'ha fatta da sola, modificando l'equilibrio unitario pensato dai costituenti del 1948. E c'è il franceschinismo di turno che invita Berlusconi a non fare riforme da solo, non tenendo conto di coloro che hanno tracciato per primi questa strada! Ma poi vi è un'altro degli aspetti più gravi della disarticolazione e della aggressione del Titolo V alla Costituzione, ed è quello che riguarda l'attacco al regionalismo unitario, che prevedeva una specialità di cinque Regioni, nella Costituzione del 1948, per ragioni di carattere storico, economico, sociale e geografico molto particolari.

perché quella riforma non soltanto ha abolito la specialità di carattere storico, ma ha inserito una doppia specialità di carattere economico, tant'è che nell'articolo 116 con quella riforma si è stabilito

parole: abbiamo una specialità di base ma, con quella riforma, le Regioni che hanno più risorse, ai sensi dell'articolo 119, possono chiedere di più allo Stato, tra le materie di competenza esclusiva dello Stato ed anche tra le materie concorrenti. Come dire che, certamente,

della Costituzione, tanto citato dalla sinistra, ove si afferma che la Repubblica si impegna ad evitare le condizioni di disuguaglianza economica, mentre con quella riforma la Repubblica protegge costituzionalmente le condizioni di ricchezza economica,

che la sinistra di Governo, sfruttando l'impazienza leghista, ha posto in essere una *devolution* dinamico-finanziaria che aveva pensato da decenni per mettere in cassaforte il proprio sistema di potere: il modello delle Regioni rosse ad alternanza zero, dove non è pensabile per l'opposizione poter vincere (e, come sappiamo, dove c'è alternanza zero non c'è democrazia, a meno di ritenere che tutti gli scienziati stiano da una parte e tutti gli imbecilli dall'altra). Ebbene, in questo contesto, di fronte ad una realtà di questo tipo, voglio dire con forza che, anche se alcuni pensano che questo sistema possa giovare alla Lega, non è così. Può darsi che Bossi lo pensi, che gli amici della Lega lo pensino. Ne dubito, anzi credo di no, perché il clima e lo sfondo sono diversi da quelli che nell'immediato dopoguerra consentirono la nascita delle Regioni rosse ad alternanza zero e la partita al Nord non è a senso unico come in Toscana o in Emilia-Romagna, ma è almeno a tre: PdL, Lega e PD, per non parlare dell'Italia dei Valori o dell'UDC. In ogni caso, a parte i dubbi sulla possibile estensione dell'alternanza zero sul piano nazionale, ritengo che dobbiamo porre presto mano alla riforma del Titolo V, perché diversamente il federalismo fiscale

al modello tosco-emiliano? Mancavano le risorse. Con questo federalismo fiscale, apparentemente non condiviso o condiviso un po' sì e un po' no, ma sostanzialmente appoggiato, la sinistra raggiunge l'obiettivo storico, quello di esistere indipendentemente dagli equilibri nazionali e dal colore politico del Governo nazionale. In questo contesto trovo veramente impressionante quello che definisco il depistaggio istituzionale di coloro che ritengono che il nostro problema sia la deriva plebiscitaria. Di fronte alla tendenza della democrazia moderna e in particolare della democrazia italiana di trasferire poteri e risorse o verso l'esterno (Comunità europea e organismi internazionali) o verso l'interno, in direzione di una molteplicità di istituzioni, di enti, di luoghi e

No! Ritengo - e lo voglio gridare con forza in questo Parlamento - che il problema non è più organizzare un assetto costituzionale contro qualcuno, come avvenuto nel 1948. Allora aveva senso perché si era in un contesto di democrazia centralista, dove poteva anche capitare che qualcuno si illudesse o comunque si desse da fare per far deragliare la giovane democrazia italiana. Ma oggi il pericolo non è più che qualcuno si impossessi di qualcosa: il pericolo è che qualcosa se ne vada per conto proprio. Oggi il nuovo assetto costituzionale deve essere pensato contro qualcosa che può disgregarsi perché si perde il riferimento unitario. Per questa ragione sostengo più *input* di sussidiarietà, di democrazia, di federalismo, ma in un contesto in cui ci siano più *input* di decisione, cioè un Parlamento forte, Regioni forti attraverso il federalismo e vicine ai cittadini e al tempo stesso un Governo forte. Solo in un contesto siffatto ritengo che si possa costruire ed avviare una nuova stagione costituente. Per tutte queste considerazioni il mio sì alla legge delega è un sì con riserva. Se si dovesse trattare dell'ultimo anello di una catena che fa saltare l'equilibrio unitario della Costituzione del 1948 evidentemente revocherò il mio sì, per quanto modesto ed insignificante, a questa legge. Ma se sarà il primo atto di una nuova stagione costituente per costruire l'Italia di domani ovviamente sarò favorevole, come sempre, a riforme che vadano in direzione della responsabilità e del coinvolgimento dei cittadini.

Resta confermato l'impianto che già il Senato aveva licenziato in prima lettura. Sono accolte positivamente la gran parte delle modifiche che la Camera ha introdotto; modifiche che hanno ancora nella gran parte dei casi migliorato e specificato il testo. Il clima costruttivo che ha accompagnato questo disegno di legge è stato confermato anche dalla discussione generale in terza lettura. Una discussione che ha visto ancora alcune differenze tra l'impostazione della maggioranza e quella dell'opposizione, ma ha visto anche un riconoscimento reciproco della bontà del lavoro svolto. Quindi ho tutta l'impressione che nel nel corso della votazione degli emendamenti le differenze rimarranno, ma altresì il reciproco riconoscimento del lavoro svolto sarà confermato. D'altra parte ho già detto, e lo confermo, che il testo oggi all'esame nella sua interezza è da noi considerato un ottimo punto di mediazione, considerato un ottimo punto di mediazione, di equilibrio e di riconoscimento della sostanza dei problemi emersi nel corso della discussione nelle Commissioni e in Aula. Dunque, credo che si possa accogliere anche la discussione di oggi come un ulteriore e positivo contributo. Penso che quando fra poco giungeremo alla discussione ed all' approvazione degli ordini del giorno si troveranno dei nuovi equilibri ancor più soddisfacenti, così da dare all' approvazione di questo testo un carattere di particolare positività. Non entro nel merito delle questioni perché già sono state più volte affrontate, lo ribadisco, in tutte le sedi possibili. I senatori hanno già mostrato nei loro interventi di conoscere bene quanto si è discusso, quanto si è approvato e quanto non si è approvato, per cui non è necessario appesantire la mia replica. Per tali ragioni,

Vorrei fare un'ultima riflessione. Il ruolo del Parlamento in questa vicenda è stato esaltato. Il Parlamento ha lavorato bene: ha introdotto una normativa su cui si è riflettuto a lungo cercando di coinvolgere tutte le energie possibili e questo è certamente un ottimo risultato;

Permettetemi di dirvi con soddisfazione che abbiamo raggiunto un buon punto di arrivo.

a partire dal relatore di minoranza Walter Vitali e tutti gli altri colleghi (che non nomino perché sono tanti), che hanno contribuito in maniera molto seria

i quattro temi che sono stati posti e che sono ancora oggetto di una possibile valutazione. Alcuni di questi li abbiamo già affrontati in Commissione, ma credo sia il caso di

Carta delle autonomie. Questa dovrebbe essere la risposta alla modifica del Titolo V del 2001 e quindi avrebbe dovuto subire un aggiornamento rispetto all'introduzione di concetti e di funzioni fondamentali trasferite o proprie,

Sono tre legislature che il Parlamento cerca inutilmente di dare queste risposte attraverso uno strumento che è sempre stato quello della legge delega

di portare non una proposta di delega, ma dispositiva. Si è deciso quindi di prendere, come si suol dire, il toro per le corna e cercare di mettere d'accordo Comuni, Province e Regioni, che fino ad oggi non hanno trovato questa intesa. Infatti, nel nuovo Titolo V abbiamo la definizione delle funzioni fondamentali (lettera *p)* del secondo comma dell'articolo 117) in capo allo Stato e alcune materie che sono contenute in quelle funzioni fondamentali oggetto, invece, di una competenza legislativa esclusiva della Regione; pertanto, questa sovrapposizione non ha portato a soluzioni condivise. Ultimamente, ancorché in via informale, abbiamo provato a fare da promotori di questi incontri per riuscire ad arrivare a scrivere le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Regioni e risolvere questa contrapposizione. Direi che sotto questo aspetto il risultato è estremamente vicino. Tuttavia, anche se è molto importante il «chi fa che cosa» - chiedo su questo un attimo di attenzione - è stato oggetto di una serie di discussioni il «quanto costa» il federalismo fiscale e se non si correrà il rischio di ulteriori duplicazioni. in maniera testarda e insistente, ho detto che tutto quello che doveva essere duplicato lo si è già realizzato. Quindi, non c'è questa possibilità. È tuttavia altrettanto evidente se si sfugge dal concetto che per una funzione non può esserci che un unico soggetto (che sia ente o altro) a detenerla o svolgerla, abbiamo fallito il nostro compito. nel momento in cui fotografo la situazione esistente, per ciascuna funzione ci sono, se va bene, tre o quattro soggetti e in alcuni casi ancora di più. Pertanto, se vogliamo che il provvedimento sul federalismo fiscale abbia una sua razionalità e una sua coerenza dobbiamo intervenire sulle duplicazioni, sulle triplicazioni, sulle quadruplicazioni, e così via.

Gruppi LNP e PdL).* Da qui la necessità di rivedere quei numeri, di considerare e promuovere l'associazionismo, perché è altrettanto evidente che un campanile, un municipio con disponibilità e cifre

che realtà di poche decine di migliaia di abitanti abbiano le municipalità piuttosto che altri soggetti e strutture che devono essere decise dal consiglio comunale? Si dice che il consiglio comunale ha poco peso:

ci sarà il problema delle Province, ma prima di operare tagli secchi voglio vedere chi fa che cosa e che cosa resta. Di alcune funzioni sono convinto, ma la mia posizione personale è che

che credo possa portare tante possibilità in più a chi amministrerà bene, chiedere una razionalizzazione degli enti locali e non vedere niente da parte dello Stato. Non mi starebbe bene:

Da tanto tempo avremmo dovuto realizzare i cosiddetti UTG (uffici territoriali del Governo) e concentrare in un unico punto tutto quello che sul territorio è rappresentato dal Governo: sono più di 96.000 dipendenti. Ha senso che questi non vengano concentrati in un unico punto a livello provinciale? A mio parere è obbligatorio farlo. Auspicherei veramente che ci fossero tanti commissari - magari i prefetti,

guardo le trasmissioni televisive, e sto meglio quando non le guardo, ma casualmente domenica sera ne ho vista una, che certo non può essere considerata filogovernativa. Ebbene, quando ho sentito parlare di strutture

di strutture con 20 posti letto e 80 medici - c'è qualcuno che magari muore perché nessuno a quel livello di territorio è in grado di eseguire un trapianto o terapie specialistiche e urgenti!

per gradi in una serie di smussature rispetto alla rigidità di tale Patto, con la necessaria e oculata resistenza anche del ministro Tremonti, il quale in questo periodo deve fare i conti con una coperta

rispetto a Comuni che hanno dimostrato la loro virtuosità quando le spese vengono destinate ad investimenti e che debba essere prevista una diversificazione.

che circolano simulazioni; se io dovessi essere virtuoso, non volendo duplicare i centri di costo, aspetterei quelle del collega Barbolini per poter risparmiare qualcosa. Il problema principale, però, è che in mezzo a tutte queste simulazioni purtroppo non c'è nulla

C'è una differenziazione completamente anomala rispetto alle previsioni di istinto, che vede una distinzione tra Est e Ovest, una diversificazione a macchia di leopardo che, sulla base di una minima analisi che abbiamo svolto, probabilmente discende da quella cristallizzazione che nel 1978 bloccò la spesa storica dei Comuni con le riforme volute da

Un metodo che mi sembra possa costituire una sperimentazione per quando andremo a parlare di Codice delle autonomie e di riforme

1a Commissione permanente, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. Esaminati i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

Colleghi, il brusìo, anche durante l'intervento del Ministro, aveva raggiunto livelli difficilmente accettabili.

specifica importanza, e vorremmo che il Governo, il relatore, ma anche i colleghi, guardassero ad esso con particolare attenzione. innanzitutto esprimere e confermare un apprezzamento per la qualità, l'intensità, nonché per l'efficacia del lavoro parlamentare che abbiamo sin qui svolto, anch'io dar atto pubblicamente al Governo, nella persona del ministro Calderoli, in primo luogo, di aver seguito con particolare attenzione e disponibilità un lavoro parlamentare così delicato.

ha qualificato l'opportunità di procedere a riforme costituzionali prescindendo da un rapporto corretto e serio di collaborazione con l'opposizione.

Ci sono però anche dei limiti in questo disegno di legge, ministro Calderoli: il limite fondamentale - non posso non sottolinearlo - è che, contrariamente a quanto l'opposizione e il Partito Democratico avevano sostenuto, il disegno di legge che giunge ad approvazione riguarda solo ed esclusivamente uno degli aspetti dell'attuazione del Titolo V della Costituzione. Si prescinde cioè da un ordine logico che avrebbe voluto - questo sì, colleghi

quali siano le funzioni dei Comuni, quali le Città metropolitane e le relative funzioni, quali le funzione residue da lasciare alle Province e quali quelle da affidare in questo contesto amministrativo alle Regioni.

che quel Titolo V, così come fu poi approvato a maggioranza, era stato votato, non solo dalla Commissione bicamerale, presieduta dall'onorevole D'Alema, con il voto favorevole del Gruppo parlamentare di cui egli faceva parte, ma di quello di tutta l'opposizione di allora:

inoltre ricordare che furono i Presidenti delle Regioni, i sindaci e i Presidenti delle Province, di ogni colore politico (da Formigoni al sindaco di Roma Rutelli), a chiedere che quello spirito costruttivo, che si era registrato nella Commissione bicamerale, si traducesse in un voto condiviso e unanime del Parlamento, per evitare che si disperdesse nella congiuntura politica così clamorosamente Francamente il ministro Calderoli, di cui ho apprezzato ancora una volta la serietà per il lavoro fin qui svolto, parlando della Carta delle autonomie poco fa ha dato prova fa ha dato prova - l'ennesima - di una certa, stravagante, eterodossia, perché egli ha illustrato le linee fondamentali della Carta delle autonomie a cui sta lavorando quasi saltando a piè pari il fatto che, se oggi non siamo nelle condizioni di approvare insieme la Carta delle autonomie con il federalismo fiscale, questo sia responsabilità di qualcun altro. Quello sforzo di semplificazione e di riduzione dei costi è uno sforzo che i senatori del Partito Democratico hanno chiesto con vigore e volevano che si realizzasse congiuntamente al federalismo fiscale. Se si è perduto tempo, signora Presidente, questo è responsabilità esclusiva del Governo, che ha perduto tempo inutilmente su questa vicenda, e dei colleghi della maggioranza, che non hanno caldeggiato con la dovuta forza l'approvazione di una rinnovata Carta delle autonomie. Ministro Calderoli, la questione degli enti locali è troppo seria per essere affrontata a colpi di *spot*; glielo dico con la consueta schiettezza e con la stima che nutro nei suoi confronti. Non si affronta la Carta delle competenze degli enti locali

Per tali ragioni, signora Presidente, noi senatori del Partito Democratico chiediamo al Governo di esprimere parere favorevole sull'ordine del giorno G100 che abbiamo presentato. Il Governo, prima in Commissione affari costituzionali con il Ministro dell'interno, poi nelle Commissioni congiunte per bocca del ministro Calderoli e del Sottosegretario, più volte ha riconfermato l'imminente presentazione di disegni di legge delega in materia di codice delle autonomie.

Chiediamo, quindi, con forza al Governo di rispettare i tempi di cui si è parlato, in modo tale che la Commissione affari costituzionali possa cominciare l'esame parlamentare del disegno di legge governativo insieme a quelli già presentati prima della pausa estiva, affinché si giunga ad una definitiva approvazione della Carta delle autonomie entro l'anno in corso. Questo, sì, darà al federalismo fiscale la forza di una riforma vera ed essenziale del Paese.

signora Presidente, che chiediamo che il Titolo V possa essere rivisto. Siamo noi - l'abbiamo sostenuto nella scorsa e in questa legislatura - a ritenere che non ha più senso

Chiediamo con forza che il Parlamento e il Governo siano disponibili ad una revisione del Titolo V della Costituzione nei termini desiderati. E, ovviamente, chiediamo che si consideri con la dovuta attenzione anche

tra finanza centrale e locale in un quadro di correzioni e contenimento della spesa che già allora contemplava un contributo rilevante degli enti locali e delle Regioni alla manovra di finanza pubblica. che si concluse un patto vero tra due contraenti e non un atto unilaterale. A quella politica di rigore, in gran parte condivisa all'epoca,

certamente il sistema delle autonomie locali non potrà sopportarla. Gli effetti delle norme restrittive sul Patto di stabilità interno, che sono certamente indotti anche dalle regole pregresse deliberate dal precedente Governo e dalla precedente maggioranza, lo sono soprattutto dalle restrizioni che ho appena indicato, di fortissimo impatto finanziario. Gli enti locali, com'è noto, dispongono di enormi risorse, di avanzi di amministrazione quantificabili in alcuni miliardi di euro che non possono spendere.

se dismettono immobili e partecipazioni non possono, contrariamente a ciò che avveniva in passato, utilizzare totalmente queste risorse per investimenti. Questi ed altri problemi poneva la mozione Franceschini, che - ricordo - è stata approvata da tutti.

alcuni di questi problemi, confinandoli all'interno di una risorsa finanziaria di 150 milioni di euro, che definire insufficiente è un eufemismo. Per dare corso agli impegni assunti dal Governo in quest'Aula e nell'altro ramo del Parlamento e solo per alleviare i problemi oggetto di quest'ordine del giorno G101 e della mozione approvata dalla Camera, occorrono alcuni miliardi di euro, non 150 milioni, altrimenti sono chiacchiere. Il ministro Tremonti, signora Presidente, ieri ha dichiarato che l'Italia starebbe affrontando meglio degli altri Paesi la crisi economica

in gran parte piccoli Comuni, che lavorano ed affrontano quotidianamente i problemi dei cittadini e delle imprese. In tutti i Paesi dell'Europa la politica economica anticrisi ha significato l'attivazione

effetti immediati sul sistema delle imprese e quindi sulla crescita. Voi, la maggioranza, questo Governo, state facendo l'esatto contrario.

previste nel Patto di stabilità per le spese di investimento dei Comuni virtuosi. C'è inoltre, sempre nel dispositivo, il riferimento ad un problema specifico, importante ed attualissimo, che riguarda il Patto di stabilità degli enti locali in Abruzzo a seguito del noto terremoto. Abbiamo letto questa mattina il testo del decreto legge sul terremoto: su questo punto e su altri - avremo modo di parlarne - è assolutamente insufficiente; occorre un impegno ‑ in questo senso va uno dei punti del dispositivo dell'ordine del giorno ‑ ad emanare una norma che riguardi tutti i Comuni colpiti dal sisma e quelli che si sono attivati per ospitare Ricordo che 40.000 persone ad oggi risiedono sulla costa come ospiti di molti Comuni che, appunto, hanno provveduto a tutto ciò cui bisognava provvedere per assistere, per far studiare i figli di quelle famiglie, per garantire i servizi e quant'altro. Vogliamo quindi impegni precisi in quest'Aula. Non si può predicare, come si è fatto fino ad oggi, il federalismo e praticare di fatto il centralismo; non si possono assumere qui in Parlamento impegni chiari e precisi e poi sistematicamente non rispettarli. I Comuni e le Province e, con essi, i cittadini e le imprese non sono mai stati così maltrattati come in questo ultimo anno, tanto da determinare la rottura dei rapporti istituzionali tra ANCI e UPI e Governo. Noi vi incalzeremo su questi punti. Chiediamo il rispetto di questi impegni questi impegni e di ribadire gli impegni stessi, che dovranno essere trasfusi in provvedimenti normativi a breve termine, non nell'interesse dei sindaci o dei Presidenti delle Province, ma nell'interesse dei cittadini, che non ce la fanno, e del sistema delle imprese, che soffre gravemente questa crisi economica.

augurandosi anche che la loro presenza aiuti i colleghi senatori ad avere un comportamento più silenzioso

di contributi ordinari, contributi consolidati e fondo sviluppo investimenti, che confluiscono nel fondo ordinario delle comunità montane. Per l'anno 2008 l'importo di questi contributi è stato determinato secondo le disposizioni della legge n. 244 del 2007, cioè la finanziaria del 2008, prevedendo rispetto al 2007 una riduzione del fondo di 30,4 milioni di euro e per l'anno 2009 di 66,8 milioni di euro. Successivamente, con il noto decreto legge n. 112 del 2008, è stata predisposta un'ulteriore riduzione dei trasferimenti erariali alle comunità montane, nella misura di 30 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. A seguito di queste riduzioni, cioè del combinato disposto delle finanziarie 2008 e 2009, si è realizzato un sostanziale azzeramento dei fondi di queste comunità. Poiché l'80 per cento del fondo è utilizzato per pagare le spese del personale, questi tagli hanno reso il fondo oggi totalmente insufficiente ad assicurare il pagamento degli stipendi e a sostenere le spese vive di funzionamento. Come lei sa, signor Presidente, le comunità montane (ad esempio della Regione Abruzzo) dall'inizio di questo mese sono nella totale e piena impossibilità di pagare gli stipendi ai propri dipendenti a tempo indeterminato, con ciò aggravando la già nota situazione di difficoltà derivante dal recente, drammatico terremoto.

ha dato alle comunità montane certezza di risorse, sulla base delle quali e nel rispetto dei limiti delle leggi sono state perseguite le politiche del personale. I tagli operati al Fondo, senza un'adeguata modifica della legislazione vigente, hanno inciso soltanto sui costi; hanno tagliato gli importi per pagare il personale, ma non hanno obbligato le Regioni ad assumere il personale. Invece, con la legislazione da noi inserita nella finanziaria del 2007, si dava a queste Regioni un tempo per realizzare questa operazione operazione di trasferimento del personale. Voi avete ulteriormente ridotto il costo, fino ad azzerarlo, ma senza dare alle Regioni l'obbligo di assumere. Una soluzione congiunturale al problema, al fine di superare l'esercizio 2009,

sia - in attesa della nuova definizione del sistema di finanza locale derivante dal varo del federalismo fiscale - in dirittura d'arrivo rispetto all'assunzione dei dipendenti che stanno attendendo. si chiede un intervento del Governo per definire la regionalizzazione dei dipendenti delle comunità montane. Le Regioni infatti, pur considerando positivamente in linea di principio la regionalizzazione del Fondo, hanno dichiarato che in questa situazione è lo Stato che deve intervenire con proprie risorse finanziarie per integrare il Fondo, a partire dalla copertura delle spese del personale in servizio presso le comunità dal 1° gennaio 2008. Con questo secondo punto il Governo si impegna ad intervenire per tutelare i dipendenti delle comunità montane, che ad oggi non hanno la certezza dell'assunzione da parte delle Regioni competenti per territorio e non possono, per loro *status*, neppure aprire un tavolo di confronto con le Regioni di appartenenza. Ora che il Governo sembra voler accogliere i contenuti di questo ordine del giorno, si dia certezza e tranquillità a quei dipendenti e alle loro famiglie, che da questo mese non percepiranno lo stipendio che loro compete.

mi appare essere molto chiaro. Questo in qualche modo mi semplifica il lavoro di illustrazione. Voglio dire in premessa che si tratta di un ordine del giorno che cerca di guardare oltre il provvedimento sul federalismo fiscale che oggi stiamo esaminando; è un ordine del giorno che cerca di compiere uno sforzo di prospettiva più ampio. Nelle premesse l'ordine del giorno ricorda che nel nostro ordinamento le riforme costituzionali, il sistema delle autonomie, le leggi elettorali e gli stessi Regolamenti parlamentari

Nel nostro ordinamento tutto deve tenersi insieme. Coerenza significa, per esempio, signor Presidente, che consistenti livelli di autonomia, con forme molto spinte di federalismo fiscale come quelle contenute nel provvedimento che stiamo esaminando, si reggono soltanto se corrispondono ad un Parlamento forte e autorevole: e non è forte, né autorevole un Parlamento eletto con liste bloccate e senza più collegi elettorali. Approvare il federalismo fiscale ci impone di riaprire subito il discorso sulla legge elettorale, qualunque sia il risultato del *referendum* che andremo a celebrare il 21 giugno. riaprire il discorso sulla legge elettorale è preliminare a qualsiasi altro discorso su altre riforme, anche di livello costituzionale. Nel dispositivo poi, l'ordine del giorno che sto illustrando impegna il Governo su tre questioni. In primo luogo, esso chiede che il Governo faccia la sua parte affinché le riforme istituzionali e quindi la nuova legge elettorale, la revisione costituzionale, i Regolamenti parlamentari

arrivammo alla modifica del Titolo V; non voglio ricordare in quale modo, molto diverso, arrivammo due legislature fa alla riforma costituzionale poi respinta

le riforme istituzionali vengano approvate su loro impegno - e l'ordine del giorno questo prevede - da una maggioranza quanto più larga possibile. Sappiamo che le riforme le approva il Parlamento, ma sappiamo anche che l'influenza politica del Governo è determinante per quel che riguarda l'orientamento della maggioranza. La seconda questione su cui l'ordine del giorno impegna impegna il Governo è a favorire una sostanziosa riduzione del numero dei parlamentari. Signor Presidente, io sono un sincero sostenitore del Parlamento

di suscitare un certo «scandalo», di ritenere che un parlamentare che faccia bene e con coscienza il suo lavoro debba essere retribuito in modo dignitoso. Non credo che, affrontando in modo demagogico il problema della

pensare che costituisca o possa costituire elemento di valutazione e selezione dei parlamentari il loro censo. Penso però che 1.000 parlamentari,

ad una corrispondente riduzione di tutti gli apparati materiali e personali oggi al servizio di Camere tanto numerose. Risparmieremmo risorse pubbliche e il Parlamento ne acquisterebbe certamente in efficienza e produttività. Il terzo ed ultimo punto su cui l'ordine del giorno che sto illustrando impegna il Governo è quello a trasformare il Senato in una Camera rappresentativa delle autonomie, ma anche e contemporaneamente - ed è un aspetto molto rilevante - a confermare il carattere unitario e indivisibile della Repubblica. Stiamo approvando una legge sul federalismo fiscale, non stiamo trasformando l'Italia da una Repubblica unitaria in una Repubblica federale e questo l'ordine del giorno chiede che venga ribadito e formalmente condiviso anche dal Governo. Chiede contemporaneamente che sia confermata la forma parlamentare e rappresentativa del nostro ordinamento costituzionale. Se dovessi giudicare dall'esperienza, dovrei concludere che l'Italia non possa rinunciare al bicameralismo perfetto. Signori senatori, se andate ad esaminare - io ho cercato di farlo farlo - il risultato del lavoro dei due rami del Parlamento nelle ultime legislature, probabilmente concludereste con me

imperfezioni che sono state sempre corrette nelle successive letture. Il bicameralismo ha finora consentito

succedere una riforma anche ordinamentale e la fine del bicameralismo perfetto per giungere ad una forma diversa di organizzazione del nostro Parlamento, nel quale una delle due Camere venga ad assumere

venga ispirata ad un lavoro responsabile che possa arrivare anche ad un livello di capacità, di efficienza politica ed istituzionale per cui la produzione legislativa sia

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono stato ben onorato e ben lieto di aver ceduto il posto nell'ordine degli interventi all'illustre senatore Zanda

Si tratta di ordini del giorno, colleghi, e non di testi di legge. Ma non vi sfugga l'importanza di questi orientamenti, perché con questi ordini del giorno tendiamo, sì, ad impegnare il Governo ma vi accorgerete bene, scorrendo il testo, che stiamo impegnando noi stessi. E alcuni autorevoli colleghi mi fanno testimonianza che quel poco che mi appresto a dirvi non lo dico adesso che ho l'onore di essere senatore, ma l'ho detto negli stessi esatti termini nella passata legislatura, quando ho avuto l'onore di essere membro della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.

giorno G103, a ben leggere, è aperto alla firma e al possibile consenso di qualunque senatore membro di questa Assemblea.

fa riferimento null'altro che alla famosa bozza della precedente legislatura (che cita in maniera numerica, quasi pudicamente,«AC

farebbe meglio a dare subito le dimissioni, in quanto esso non solo certifica l'inutilità del Senato, ma addirittura proclama che esso è un inutile e dannoso impaccio al procedimento legislativo. Che questo lo faccia la Camera dei deputati non trova certo spazio di elogio; tuttavia lo si può pur comprendere. Se però lo facesse il Senato sarebbe un momento di interlocuzione al ribasso che francamente mi lascerebbe sconcertato. Ci saranno momenti di interlocuzione nell'*iter* più o meno lungo delle riforme istituzionali, ma che il Senato della Repubblica parta in questo processo di interlocuzione con l'affermazione della propria inutilità e dell'opportunità della propria cancellazione come Camera parlamentare è cosa che sbalordirebbe noi stessi e l'opinione pubblica. Ve lo dice chi è stato onorato dalla partecipazione a quattro legislature della Camera e che - parlano i verbali, oltre agli autorevoli testimoni che ho citato prima - ha detto le stesse cose un anno fa a Montecitorio, quando neppure pensava di avere l'onore di venire in Senato.

ne richiama i contenuti. È dunque dettagliatissimo. Chi dei senatori non sa che quella bozza prevede il superamento del bicameralismo perfetto in un modo molto semplice? La Camera resta tal quale, organo deliberante politico e sovrano eletto dal popolo, il Senato si riduce. Non capisco poi perché lo chiamino ancora con il pomposo nome di Senato federale della Repubblica, quando la *senectus* non c'è più (perché i suoi membri quando ha poteri deliberativi eventuali e subordinati (con 30 firme ha facoltà di richiamare un testo per dare suggerimenti alla Camera, la quale poi però delibera definitivamente, tenendone o non tenendone conto, per quasi tutte le leggi, eccetto quelle di rilievo costituzionale, dove è previsto il voto congiunto). Quanto poi alle modalità di composizione e di elezione non sarebbe altro che un'assembleina di 180‑200 delegati, consiglieri regionali, provinciali e comunali, che restano tali in carica e che a, mezzo servizio, fanno i cosiddetti senatori. Non capisco l'orpello di questo nome così sontuoso

che non potrei che liquidarlo dicendo: «Forse tu dici il contrario perché stai vegetando alla Camera». Non mi abbasso a questo, ma dico che con il mio ordine del giorno, trattabile e confrontabile (nel mentre respingo risolutamente ed invito l'Aula tutta,

dicevo, al rafforzamento dei poteri del Premier, alla previsione della cosiddetta regola della sfiducia costruttiva ed alla ragionevole, collega Zanda, diminuzione del numero dei parlamentari di entrambi i rami.

E poi, rovesciando i termini del problema, prefiguro - non certo disciplinando - un Senato della Repubblica come Camera Alta, luogo della rappresentanza del pluralismo politico democratico, che ha il voto di fiducia nei confronti dell'Esecutivo e che dà l'ultima deliberazione, mantenendo il bicameralismo pieno a questo riguardo sulle leggi all'esame del Parlamento. Concepisco, prefiguro e ipotizzo una Camera dei deputati o dei rappresentanti come Camera Bassa, con la «b» maiuscola, come luogo della rappresentanza del pluralismo territoriale e sociale, che non si esaurisce cioè nel mero pluralismo politico, che concorre anch'essa all'esame, al varo, al voto delle leggi, seppure avendo il Senato della Repubblica - o Camera Alta, se preferite - il voto definitivo. G103 non cancella l'ipotesi del bicameralismo, ma supera il bicameralismo perfetto, concependo due Camere ugualmente investite di potere sovrano democratico, elette direttamente dal popolo, ma con un ruolo parzialmente diverso. A mio personalissimo modo di vedere, onorevoli senatori, ove si dovesse concepire una differenziazione diversa, dovrei solo poter concepire in questo momento un Senato (Camera Alta, sempre) che si occupi degli aspetti di rilievo costituzionale, una sorta di Commissione affari costituzionali eretta a Camera parlamentare. Potrei concepire questo; in qualche Paese esiste, in qualche altro Paese esiste qualche cosa che è la caricatura di quella che sarebbe la bozza di cui ci stiamo occupando e le delegazioni estere, che ci hanno fatto visita, ci hanno spiegato le gravi incongruenze a cui stanno andando incontro. Questa è l'illustrazione a braccio, ma credo abbastanza chiara, dell'ordine del giorno a mia firma, che non è dunque una mera rivendicazione di esistenza, perché tutto questo avvilirebbe addirittura il profilo culturale del nostro dibattito. Esso, invece, richiama all'attenzione dei nostri colleghi parlamentari l'opportunità e la necessità che, mentre licenziamo una riforma così importante come è il federalismo fiscale - e tutti riconosciamo essere necessario che ad esso seguano e siano complementari riforme istituzionali di grande rilievo - si proceda, quanto più possibile con un consenso ampio tra maggioranza e opposizione e con la sintonia del Governo con l'opposizione, non meno che con la sua maggioranza (che finalmente dovrà essere anch'essa consultata, fino a prova contraria), e si possa arrivare a questo tipo di riforme. Si tratta pertanto di una proposta costruttiva; anche sui documenti, io e gli altri 50 o 60 onorevoli senatori che mi hanno onorato della loro firma siamo pronti naturalmente a soprassedere al voto, a confrontarci, a vedere se si può arrivare ad un testo unitario, che conservi però il principio che il bicameralismo perfetto si può superare solo con la preservazione di una dignità e di una pienezza di poteri parlamentari fondata e giustificata sull'investitura diretta del popolo e sulla differenziazione della conformazione e delle risorse operative e deliberative delle due Camere. Questo con tutta franchezza mi sembra, senza retropensieri, senza tatticismi di alcun genere - che mi sono assolutamente odiosi oltre che molesti il nostro pensiero (non dico solo il mio, ma di numerosi membri della maggioranza parlamentare), sul quale mi auguro si possa fare senza fretta - perché su argomenti di questo genere la fretta sarebbe colpevole e cattiva consigliera - un confronto costruttivo per ogni possibilità di incontro sulle rispettive tesi.

per gli ordini del giorno dobbiamo arrivare a puntuali riformulazioni - alcune già concordate, altre da perfezionare

scorso dalla Camera; a prevedere, una verifica, da espletare entro il 30 giugno, degli effetti che le norme in vigore hanno prodotto sull'andamento complessivo dei saldi di finanza pubblica, ai fini di un aggiornamento delle norme sul Patto di stabilità interno per le spese di investimento dei comuni virtuosi; a prevedere

tutti gli enti locali colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo».

Presidente, con i numerosi colleghi firmatari ci accomoderemmo a mutilare l'ordine del giorno salvandone, in definitiva, due soli punti purché,

Signor Presidente, il Partito Democratico ha seguito i lavori su questo provvedimento con uno spirito costruttivo evidente. Non si è trattato soltanto della più totale assenza di qualsiasi intervento di carattere ostruzionistico, ma siamo intervenuti nella prima e nella seconda lettura contribuendo, a mio parere, in modo decisivo a un consistente miglioramento del provvedimento. Abbiamo adottato lo stesso metodo di lavoro anche per quanto riguarda

discutere insieme quali possibilità vi fossero per arrivare a ordini del giorno condivisi da Governo, relatore e presentatori. Sull'ordine del giorno G104, di cui sono primo firmatario, abbiamo raggiunto un'intesa. Il Governo e il relatore hanno proposto una modifica e il Governo mi ha fatto pervenire questa modifica

Voglio rilevare - lo dico senza spirito polemico - che c'è stato un tempo nel quale si potevano rimettere a posto gli orologi sulla scansione del tempo dei lavori del Senato. La seduta è rimasta sospesa, come lei stesso ha giustamente rilevato, per quasi 15 minuti ed è ripresa soltanto perché lei è intervenuto in modo consistente. Adesso mi viene proposta in Aula un'ulteriore modifica che considero assolutamente immotivata e che contrasta con l'accordo raggiunto questa stessa mattina con il Governo e con il relatore. Non posso accettare questa modifica.

il Governo rispetto a posizioni che saranno squisitamente parlamentari e delle Assemblee rispetto alla struttura stessa del Parlamento.

non credo che debba esserci oggi una competizione tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica nell'attribuirsi la qualifica di Camera alta piuttosto che bassa e che si debba fare quasi uno scontro bicamerale e non un concorso. Mi sembra che quello che sta emergendo - e non vorrei mai che fosse così perché altrimenti le riforme non le faremmo mai - è il timore che il Senato diventi una Camera di serie B rispetto alla Camera dei deputati. Cambierà la sua natura e farà qualcosa di diverso, ma ritengo che quel qualcosa di diverso sarà tale per cui il rilievo istituzionale del Senato potrà mettere addirittura in difficoltà la Camera che esprime la fiducia, perché comunque i passaggi di cui si occuperà il Senato rispetto agli *iter* legislativi,

ai senatori dei *Länder* il rilievo e il peso che hanno all'interno del sistema federale tedesco! Se partiamo da questo principio,

Personalmente non ritengo - è una mia impressione personale - che debba o possa essere l'ordine del giorno in quanto tale, come strumento,

se intendesse coinvolgere e informare i cittadini, i comitati e gli enti locali interessati sullo stato di avanzamento del progetto di stoccaggio del gas a Rivara di San Felice, un Comune del modenese, e sull'istanza presentata dalla Società Indipendent Gas Management per la realizzazione del sito di stoccaggio, nonché delle relative procedure di valutazione di merito. La richiesta di sollecitazione è legata al fatto che il 24 aprile scorso, a seguito di un incontro che si è tenuto a Rivara, il vice presidente nazionale del CODACONS

conoscenze che non può esplicitare in un'assemblea pubblica, e che hanno gettato in uno stato di tensione i cittadini, oppure il Governo non può sottrarsi alle procedure previste, compresa l'espressione preliminare della commissione VIA e soprattutto il coinvolgimento, nella

Signora Presidente, il 2 maggio il ministro Rotondi sarà ad Alessandria per incontrare la comunità piemontese per una verifica degli impegni del Governo. Proprio in queste ore 6.000 cittadini sono stati evacuati da Alessandria per la piena del Tanaro.

ha già prodotto 5.600 milioni di euro dovuti alla Regione Piemonte, parte dei quali potrebbero essere utilizzati per mettere in sicurezza il territorio. i fondi regionali della Protezione civile sono stati tagliati e non è stato possibile in finanziaria trovare le risorse necessarie per la messa in sicurezza di un territorio che parte dal Piemonte, ma si estende per tutta l'asta del tutta l'asta del fiume Po, che in questi giorni è coinvolta da esondazioni significative. È quindi importante, e lo dico in modo che il ministro Rotondi lo sappia prima, che la legge n. 35 del 1995 veda almeno una parziale attuazione: adesso c'è il bisogno, adesso ci sono le risorse, adesso possiamo in parte colmare l'impossibilità che il Governo ha dimostrato in sede di finanziaria e nelle discussioni successive. Signora Presidente, questa legislatura compie oggi il suo primo anno di vita; è tempo dunque di bilanci ed un bilancio mi sembra meriti un

la sobrietà e l'attenzione a problemi cruciali e quindi scartando tutte le sollecitazioni per interrogazioni di carattere opportunistico o comunque relative a problemi di dettaglio, ho presentato otto interrogazioni,

un'interrogazione al Presidente, per sapere se egli non ritenga che questo comportamento del Governo abbia l'effetto di azzerare una prerogativa costituzionale del Parlamento, alterando il rapporto istituito dalla Carta tra i due organi, organi, Governo e Parlamento; conseguentemente, far sapere se il Presidente non ritenga di intervenire in modo severo e rigoroso nei confronti del Governo per esigere che esso cessi di sottrarsi sistematicamente al sindacato ispettivo del Parlamento.